In data 19 settembre scorso, da parte del direttore del Consiglio italiano per i rifugiati, Christopher Hein, è stata inviata una lettera al sottosegretario di Stato per l'interno Lucidi, con la quale si esprimono le doglianze di questa associazione perché i respingimenti e le espulsioni sono troppo numerosi dai porti di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Signor Presidente, a parte il discorso che sentiamo in questi giorni a proposito dell'emergenza criminalità e dell'emergenza rappresentata da tutti questi ingressi, la cosa sorprendente è che da quando è arrivata questa lettera evidentemente è stata data qualche disposizione e da allora si sono bloccati tutti i respingimenti. Le faccio presente anche che su «Il Gazzettino» di oggi c'è scritto: «Emergenza romeni: a Nordest zero espulsioni». Vorrei che il Governo venisse in Aula per rispondere a questa

relativamente alla scomparsa, che annuncio all'Assemblea, del giornalista Enzo Biagi, che, come sapete, è stato un grande giornalista italiano, un grande storico italiano, un «giornalista libero», come l'ha definito il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La Presidenza ritiene di dover dare la parola a chi l'ha chiesta. Vi pregherei però di tener conto che ci sono degli adempimenti che dobbiamo svolgere riguardanti il nostro lavoro, a cui ha fatto riferimento ieri il Presidente. Darò quindi la parola a chi l'ha chiesta per non più di un minuto

Presidente, con Enzo Biagi viene a mancare non solo un grande giornalista, ma anche un uomo che con il suo impegno civile

diffusi, soprattutto in quella parte di lettori che amava certe rievocazioni di Enzo Biagi, che rimangono scolpite nella nostra memoria

che ha avuto per l'Italia e per i giovani italiani una funzione straordinariamente pedagogica. La capacità della resa in parole semplici non soltanto della verità, così come Biagi grande giornalista riusciva a vedere e a descrivere,

mi fa piacere che questa richiesta di ricordo venga anche dei banchi dell'opposizione. Credo che in questo senso Enzo Biagi appartenga alla migliore tradizione del giornalismo italiano, alla migliore tradizione

partigiano di giustizia e libertà. Rimase per tutta la vita fedele ad una scelta di socialismo umanitario che lo caratterizzò, senza enfasi, senza rigidità e con grande apertura anche ad esperienze o ad afflati religiosi non schierati e clericali intensi e profondi. Credo che sia questa la cifra storica con cui questo grande personaggio rimane tra noi nella memoria. In particolare, voglio ricordare tra le sue tantissime produzioni gli ultimi programmi che presentò in televisione, che furono soprattutto il segno che aveva ricostruito una redazione piena di giovani ai quali non voleva ostacolare la carriera. Due grandi insegnamenti di contenuto personale, di fedeltà a se stesso senza rigidità e anche di apertura non egoistica agli altri, doti rarissime nel mondo giornalistico, per non dire in quello politico. *(Applausi

Il momento di questa mattina è particolarmente emozionante per quelli di noi - ed è il mio caso che hanno lavorato per una vita accanto ad Enzo Biagi, condividendo per una vita il modo in cui Enzo Biagi è stato giornalista. Una commemorazione, un ricordo di Enzo Biagi, non può essere fazioso perché lui non è mai stato tale: è stato, invero, un testimone, ha interpretato il giornalismo come testimonianza

tutto fatti, tutto accertamento della realtà. La parola "verità" non gli si addice perché verità si scrive troppo spesso con la "v" maiuscola. La parola "realtà" era la sua parola: lavorando con lui ed accanto a lui abbiamo imparato quanta dignità possa avere il mestiere di giornalista; una dignità che senza Enzo Biagi un po' si disperde. *(Applausi dal Signor Presidente, anche noi ci associamo a questo ricordo in una giornata in cui il giornalismo italiano ha perso un grande personaggio. Quando

di un Paese. Enzo Biagi ha, con le sue opinioni, contribuito a questo e di ciò gli siamo grati. con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani rende omaggio alla figura di Enzo Biagi: una figura luminosa di giornalista, di scrittore, di divulgatore; di uomo libero che si è impegnato a difendere la libertà di tutti.

un grande giornalista che ha accompagnato tanta parte della nostra vita, della nostra attività, delle nostre vicende, aiutandoci a comprendere con semplicità e con mente liberale le vicende politiche e la storia dell'Italia, soprattutto avendo la capacità di trasmettere ai giovani il valore della nostra storia. Oltre al cordoglio umano per un'esistenza che si è conclusa in serenità, ci mancherà soprattutto quella sua ineguagliabile capacità di estrarre dai fatti, anche i più minuti, il senso profondo della storia e della società italiana.

nelle parole, nel raccontare i fatti, nel ragionare, nel richiedere ed interrogare la realtà di un giornalista così importante che, come altri hanno ricordato, è stato un punto di riferimento ed ha costruito con noi

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che, a prescindere dalle rappresentazioni a tinte accese che della situazione politica generale, particolarmente del clima di *suspense* che ci sarebbe in questa Aula in concomitanza con il passaggio della finanziaria 2007, vengono date al Paese ogni giorno dalla televisione e dalla stampa, nonostante queste rappresentazioni ad effetto, il clima parlamentare e sociale di oggi sia assai meno teso di quello che caratterizzò la discussione parlamentare della finanziaria 2007. Indubbiamente, oggi avvertiamo il peso di una maggioranza già estremamente risicata in base al risultato elettorale e che si è ulteriormente indebolita, in qualche caso per ragioni personalistiche, più spesso anche per oggettive differenziazioni di sensibilità e di approccio ai problemi tra le diverse forze che compongono uno schieramento tanto politicamente composito. Proprio la crudezza dei dati di partenza, cioè l'esiguità ontologica della maggioranza in questa Aula e la situazione economica che fu necessario affrontare subito nel 2006 con la manovra correttiva e la finanziaria 2007, complessivamente per oltre 40 miliardi di euro, dovrebbe suscitare grande apprezzamento per una generosa e complessa azione di Governo, che, nonostante tutto, riesce comunque a trasformarsi, dapprima in provvedimenti di legge e successivamente in risanamento finanziario, in azione di sviluppo, in equità sociale, in modernizzazione dell'apparato istituzionale e liberalizzazione dei processi economici. Tenendo conto di questo stato di cose, c'è da ritenere che alcuni dei risultati realizzati siano addirittura eccezionali, come anche è singolare il fatto che di essi i *media* e l'opinione pubblica non siano sufficientemente avvertiti. Dall'inizio della legislatura, infatti, si è registrata la riduzione dell'indebitamento netto, passato dal 4,4 per cento del PIL nel 2006, cento nel 2007; per il 2008 esso si ridurrà ulteriormente sino al 2,2 per cento. L'andamento del debito pubblico è decrescente e raggiungerà il valore del 103,5 per cento del PIL nel 2008. L'avanzo primario, dopo essere stato azzerato negli anni passati, si attesterà al 2,6 per cento nel 2008. La politica economica del Governo ha dunque privilegiato l'individuazione di un equilibrio tra misure di risanamento, di impulso allo sviluppo, di attenuazione della pressione fiscale e di riduzione delle disuguaglianze sociali. La manovra finanziaria per il 2008 ha l'obiettivo di proseguire nella realizzazione dell'equilibrio finanziario, volto a contemperare le esigenze di risanamento, di crescita economica, di equità, nonché di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione, anche attraverso una maggiore trasparenza del bilancio dello Stato. Sul tema del Mezzogiorno l'azione del bilancio 2008 si caratterizza non solo per i nuovi finanziamenti, ma anche e soprattutto per il più efficace utilizzo delle risorse disponibili. Le nuove risorse connesse all'attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013 in cui vengono fatti confluire il fondo per le aree sottoutilizzate ed i fondi europei, ammontanti ad oltre 100 miliardi di euro, rappresentano un'occasione importante per ammodernare e potenziare le infrastrutture del Paese e recuperare il Mezzogiorno all'economia produttiva, consentendo anche al sistema economico nazionale di colmare il ritardo di competitività e di crescita rispetto ai principali Paesi europei. In un quadro economico caratterizzato dal contenimento della spesa, la manovra di bilancio propone risorse aggiuntive per oltre 200 milioni di euro per il comparto della sicurezza. Per la giustizia è di particolare rilievo l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, circa 70 milioni nel prossimo triennio, volto a fronteggiare situazioni di emergenza in questo settore con l'adeguamento strutturale degli edifici esistenti, oltre che con la realizzazione di nuove strutture. Si apprezzano inoltre le previsioni che autorizzano per l'anno in corso la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione della banca dati delle misure cautelari, oltre che il rafforzamento della struttura informatica del registro generale del casellario giudiziario e la sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione. A questo proposito, desidero tuttavia rimarcare la prioritaria necessità di un finanziamento adeguato delle operazioni di digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, compresi l'aggiornamento informatico del casellario giudiziario nonché dei processi civili e penali. Si avvierebbe, infatti, un'evidente razionalizzazione delle risorse, connessa all'aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della giustizia nel suo complesso. Gli investimenti informatici si dimostrano infatti, almeno nel lungo periodo, altamente redditizi perché consentono la realizzazione di numerose economie di scala. Tra le altre misure contenute nel testo della manovra, desidero evidenziare le disposizioni tributarie volte alla riforma dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che vanno nel senso di assicurare una complessiva semplificazione e riduzione del peso delle imposte e, conseguentemente, di favorire la competitività del sistema imprenditoriale. Gli interventi nel settore tributario perseguono le già richiamate finalità di sviluppo e di equità, come ad esempio le disposizioni tese ad introdurre un regime fiscale *ad hoc* per le imprese minime e marginali, nonché altre misure in favore delle imprese, tra cui il rafforzamento del credito d'imposta per la ricerca e la ridefinizione del fondo per la finanza d'impresa. La finanziaria ha anche un particolare riguardo alle politiche sociali, alle politiche per la casa, con un riferimento alla riduzione del carico fiscale riguardante l'imposta comunale sugli immobili, sulle abitazioni di residenza dei proprietari, la concessione di agevolazioni fiscali per le locazioni degli immobili, l'introduzione di deduzioni IRPEF sulla prima casa, il rilancio delle politiche abitative per i ceti sociali meno abbienti e le giovani coppie, la conferma delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici nonché la proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Si segnalano inoltre significativi aumenti degli investimenti infrastrutturali e il miglioramento della sicurezza del sistema dei trasporti nazionali e locali, nel quadro di una rinnovata attenzione nei confronti delle modalità con un minore impatto ambientale. Al riguardo, ricordo l'istituzione del fondo per la mobilità locale, destinato al miglioramento del trasporto pubblico, l'agevolazione fiscale per gli abbonamenti ai servizi di trasporto locale, nonché le iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intermodalità, alla diversificazione dei mezzi di trasporto e all'innalzamento della quantità e del livello dei servizi. La legge finanziaria per il 2008 ha per il sistema delle autonomie locali un merito, che costituisce la base di partenza per qualsiasi analisi, osservazione e giudizio di valore sulle singole disposizioni:

Le modifiche apportate al Patto di stabilità interno, coerentemente con gli impegni presi dal Governo, rendono il sistema più aderente a quello europeo, riconoscendo maggiore discrezionalità ai Comuni nella gestione dei flussi finanziari, e rappresentano un netto miglioramento rispetto alla finanziaria dello scorso anno. In riferimento al tema dell'equità, la manovra di bilancio, con i provvedimenti che l'hanno preceduta, contiene una fitta rete di interventi su una pluralità di settori cruciali per la vita della nostra società; per i soggetti con redditi inferiori al minimo imponibile, un *bonus* di nuova ideazione assicurerà un aiuto concreto, anche se limitato, in tempi brevi; s'introduce il congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento, effettuando una completa equiparazione a quanto previsto per i figli biologici. Vengono estesi anche i benefìci riconosciuti alle vittime del terrorismo e del crimine nonché ai loro familiari superstiti. Prosegue la politica di contrasto della violenza alle donne con un incremento significativo dei fondi destinati a questo scopo. Si introduce uno sconto fiscale ai giovani tra i 20 e i 30 anni che affittano casa e viene ampliato lo sconto per le locazioni degli studenti universitari. In tema di lavoro, lo sforzo si è applicato ad accrescere l'efficacia della disciplina del mercato, ad incoraggiare una partecipazione sempre più alta alle forze di lavoro e ad offrire tutele adeguate contro il rischio di percorsi lavorativi frammentati. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una finanziaria snella, trasparente e leggibile, frutto di cooperazione con e tra le principali istituzioni e rappresentanze del Paese. Accoglie il risultato di accordi ed intese con il sistema delle autonomie locali, con le parti sociali e con i rappresentanti di numerosissimi settori della vita civile ed economica del Paese. Questa finanziaria ha l'ambizione di farci tornare a crescere per dare una prospettiva ai giovani, per incrementare i livelli di benessere, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, l'influenza internazionale e le giuste ambizioni, cioè, di un Paese industriale avanzato. Proprio questi dati mi inducono a ritenere che il Governo, pur con tutti i problemi della maggioranza che lo sorregge, abbia meriti importanti, uno in particolare: non guarda ai problemi del Paese con l'ansia del consenso immediato; se avesse voluto questo, già nel 2006 avrebbe fatto una finanziaria da 20 miliardi di euro. In una società come quella italiana, frammentata, contraddittoria, poco incline al rispetto delle regole, con un sistema istituzionale poco adatto a decidere, il Governo ha dimostrato di saper operare per sintesi, individuando le priorità che veramente potranno garantire il Paese nei tempi medio lunghi. D'altro canto, questo Governo viene accusato di tutto: di mettere molte tasse ma anche di ridurle senza idonea copertura, di comprimere i redditi ma anche di avere predisposto una finanza assistenziale pensata con logica elettorale. Forse sono critiche giustificate, ma forse è proprio questa la politica che predichiamo da molto tempo. Non possono esserci due tempi diversi tra il risanamento finanziario e il sostegno a chi è in difficoltà. E poi perché deve essere il solo Governatore della Banca d'Italia a rappresentare la necessità che i redditi di lavoro aumentino e che venga ridotta l'area della precarietà? È bene che queste cose le dica il governatore Draghi, ma è assai più giusto e normale che queste cose le dica e le faccia la politica, e in particolare una maggioranza di centro-sinistra. I fatti sono ostinati e la loro forza alla fine sarà irresistibile.

brevemente sulla rilevanza della riforma delle energie rinnovabili per produrre energia elettrica, riforma introdotta con alcuni articoli aggiuntivi (30-*bis* e successivi) dalla Commissione bilancio nel disegno di legge finanziaria al nostro esame. In particolare, intervengo per evidenziare non solo la rilevanza ambientale di tale provvedimento, ma anche la sua portata economica sul sistema energetico ed economico del Paese. L'Unione Europea, nel marzo 2007, con documento del Consiglio ha varato alcuni obiettivi ambiziosi che, per la prima volta, sono indicati come obiettivi vincolanti per i Paesi dell'Unione Europea. Fra questi obiettivi rientra il 20 per cento di fonti rinnovabili - il 20 per cento è il consumo lordo dell'Unione europea - da raggiungere entro il 2020. Questo richiede innanzitutto un nuovo e più vigoroso impegno di tutti i Paesi dell'Unione nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2000, nell'Unione europea, era di circa 400 terawattora ed è passata nel 2005 a 463 terawattora. un incremento significativo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei 25 Paesi dell'Unione Europea di oltre 60 terawattora nei cinque anni che vanno dal 2000 al 2005. La Germania ha guidato questa

il quesito al quale questa riforma dà una risposta. La risposta non è che il sistema di incentivazione era meno generoso in Italia che in Europa. risposta è che una quota consistente di questa incentivazione è stata impropriamente destinata, attraverso il CIP6, a fonti non rinnovabili attraverso le cosiddette fonti assimilate.

al nostro sistema di incentivazione non ha prodotto rilevanti risultati, visto che la produzione in terawattora è rimasta sostanzialmente ferma negli ultimi cinque anni. La riforma promossa da questi articoli aggiuntivi innanzitutto modifica il sistema di incentivazione,

Un sistema di tariffa fissa consente infatti di dare certezza agli investimenti e ciò è vero, a maggior ragione, se questa tariffa è differenziata sulla base della fonte. i costi di produzione non sono uguali su tutte le fonti rinnovabili e, avendo il certificato verde nel vecchio sistema lo stesso valore, esso rischiava di incentivare troppo fonti più mature e troppo poco fonti non ancora mature.

Il certificato verde di un megawatt ora è portato a 180 euro al megawattora, cioè a 18 centesimi di euro.

l'incentivazione complessiva sulle fonti energetiche rinnovabili: prolungando però la durata del certificato verde a 15 anni per tutti si consente di distribuire questo vantaggio rispetto agli 8 anni di partenza e ai 12 intermedi introdotti su un maggior numero di anni, garantendo quindi agli investitori vantaggi equivalenti ed ottenendo però una migliore distribuzione sulla tariffa elettrica. La riforma produce importanti effetti. Tra l'altro, recupera anche un tema che non rendeva efficace l'anticipo di questa riforma che abbiamo approvato nel decreto fiscale collegato alla finanziaria per le biomasse da contratto di filiera e da filiera corta ovviamente di origine agricola, le quali biomasse

di tale sistema, che intanto avviene in contemporanea col taglio del CIP6 per le fonti non rinnovabili, che consentirà un risparmio entro il 2012 di 1,3 miliardi di euro, che potranno essere ben utilizzati nell'incentivazione delle fonti rinnovabili. Inoltre, questo sistema a regime produrrà un risparmio di emissioni di CO2 di circa 30 milioni di tonnellate, che moltiplicate per il costo di tonnellate della CO2 produrrà un risparmio di 750 milioni di euro all'anno. Infine, vi è il vantaggio nella riduzione delle importazioni di petrolio o comunque nella dipendenza energetica del Paese:

di una riforma importante, che avrà un impatto economico significativo e positivo sulla competitività del Paese, e sul sistema energetico nel suo complesso. *(Applausi del senatore Ferrante)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

Cosa si è fatto, di concreto, in questa finanziaria per il rilancio dell'economia, soprattutto nei settori altamente innovativi che dovrebbero fare da traino nel futuro del nostro Pese? Pese? Prendo ad esempio il settore farmaceutico, materia di competenza della Commissione di cui faccio parte. Tutti sappiamo che l'industria farmaceutica è unanimemente ritenuta come uno dei settori strategici che dovrebbero consentire anche all'Italia di allinearsi agli altri principali *partner* europei nel finalizzare quanto prefissatosi in occasione degli incontri di Lisbona e Barcellona, ovvero investimenti in ricerca e sviluppo pari al 3 per cento del PIL entro il 2010 (ricordo che oggi l'Italia è di poco sopra all'uno con un *trend* addirittura in calo negli ultimi anni). Il farmaceutico è infatti un settore che vede in Italia ben 8 ricercatori su 100 occupati, rispetto ad una media dell'industria manifatturiera che è di un ricercatore ogni 100 occupati. È un settore molto importante per la nostra economia. Le esportazioni di farmaci hanno raggiunto i 9,3 miliardi di euro, i dipendenti sono 74.000 di cui circa 6.200 ricercatori, più altri 240.000 addetti nell'indotto.

Rispetto ai 6.200 ricercatori italiani, ve ne sono più di 22.000 in Francia, 21.000 nel Regno Unito, 15.300 in Germania. A fronte del miliardo di euro annuo investito in ricerca e sviluppo in Italia, ne abbiamo 4,8 nel Regno Unito, 4,0 in Francia e 3,9 in Germania. Ed è subito fatto il conto, colleghi. Ai nostri 9,3 miliardi di euro in *export* corrispondono i circa 26 della Germania, 17,5 del Regno Unito e i 16,5 della Francia. Occorre quindi liberare le enormi potenzialità di crescita del settore, togliendo gli ostacoli che ad oggi ne hanno rappresentato un freno allo sviluppo. Tale posizione mi pare sia ampiamente condivisa anche all'interno della maggioranza,

Il Governo intende dunque correggere le distorsioni e creare le condizioni per ricominciare ad attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e nelle attività produttive» e che «è inutile nascondere che il mercato farmaceutico italiano e le sue regole siano state influenzate più dalle politiche pubbliche di natura macroeconomica che da quelle industriali di settore. Questa anomalia va corretta». È evidente È evidente che per incoraggiare gli investimenti occorrono prezzi remunerativi, e la sicurezza che il frutto della ricerca sia adeguatamente protetto dal brevetto. Per quanto riguarda la situazione prezzi, l'Italia si trova ai livelli più bassi d'Europa, come testimoniato da uno studio uscito in questi giorni e prodotto dal CERGAS, istituto dell'Università Bocconi di Milano, con differenze per i prodotti di più recente commercializzazione mediamente del 20 per cento, con punte anche del - 40 Per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti derivanti dal brevetto, nel corso dell'anno 2006 molte Regioni hanno introdotto (al momento nella classe degli antiulcera) il meccanismo di rimborso denominato *reference price*, che coinvolge anche i prodotti coperti da brevetto: da brevetto: il prezzo rimborsato al cittadino è quello del prodotto a prezzo più basso e ormai con il brevetto scaduto, per cui tutti gli altri prodotti della classe o si allineano a quel prezzo, o perdono in pratica la quasi totalità delle vendite. Ovviamente, i prodotti non più coperti da brevetto hanno ormai ammortizzato gli investimenti in ricerca e quindi possono ridurre il prezzo anche del 50 per cento rispetto agli altri prodotti. prodotti. Con questo meccanismo l'azienda non si trova più nelle condizioni di avere la certezza dei diritti derivati della copertura brevettale e quindi - purtroppo questo è il grosso problema - non ha più la possibilità di recuperare gli investimenti fatti in ricerca. Questo è un fattore determinante per scoraggiare qualsiasi investimento in tal senso. Cosa è contenuto ad oggi nella finanziaria 2008 su questi due importantissimi aspetti, che oggettivamente rappresentano un enorme ostacolo allo sviluppo del settore? Sul fronte prezzi nessuna novità è stata introdotta, se non un meccanismo estremamente dirigistico di *budget* aziendali, che oltre a congelare i prezzi al livello attuale, di fatto introduce delle forti limitazioni alla naturale dinamica concorrenziale, bloccando le quote di mercato delle aziende e la loro possibilità di sviluppo. Viene oltretutto inserita la brillante - in senso ironico - novità del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutico addossato interamente al settore privato (quando fino ad oggi concorrono le Regioni per un 40 per cento) per le vendite in farmacia, circostanza che porterebbe alla situazione assurda che le aziende si troverebbero a dover restituire interamente quanto incassato dalla vendite di questi prodotti, con l'impossibilità quindi di coprire almeno in parte i costi sostenuti. Molte altre sono le contraddizioni presenti: per esempio, i prodotti cosiddetti innovativi di nuova immissione in commercio sfondano il loro *budget*, ripianano gli altri prodotti ma non i vecchi farmaci con il brevetto scaduto. Per quanto riguarda poi l'abolizione del *reference price*, sempre ad oggi questa opzione non è prevista nel testo della legge. Spero vivamente che almeno su questi due aspetti il Governo voglia apportare le necessarie modifiche almeno in questo caso, ci sia un seguito tra quello che si dice e quello che si fa, ovvero dare impulso ai settori strategici e nella fattispecie a quello farmaceutico. Se però anche in questo caso il Governo non intende porsi il problema, allora è meglio, cari colleghi, che vada a casa e lasci spazio a chi ha dimostrato di saper lavorare garantendo la ricerca e l'occupazione. *(Applausi dal

Non sarebbe auspicabile perciò che, nei rivoli della polemica di queste ore, si perdesse il dato qualificante di questo disegno generale: non una legge *omnibus* di norme e interventi ordinamentali, ma la destinazione delle risorse dello Stato, in modo leggibile e chiaro, a favore dei cittadini. È una finanziaria seria, che non mette le mani nelle tasche degli italiani, ma restituisce e aiuta i più deboli. E questo non è frutto solo di una chiara volontà politica, ma anche e soprattutto delle condizioni che, faticosamente, il centro-sinistra ha creato nel corso di quest'anno. In diciotto mesi, con due decreti, sono stati restituiti ai cittadini più di 13 miliardi di euro e oggi possiamo affrontare con serenità una finanziaria che riduce il peso fiscale per i lavoratori, per i cittadini, per le imprese. Tutto questo è frutto del serrato e compatto impegno della nostra maggioranza contro l'evasione fiscale. La scelta ferma di fare del recupero di quei 200 miliardi rubati al fisco il primo dei nostri obiettivi ci consente, con serietà, di avviare un grande intervento di redistribuzione. E questo impegno, come dimostra la scelta di rafforzare l'Agenzia delle entrate con nuovo personale, proseguirà con decisione. Non si tratta solo di recuperare risorse sottratte alla collettività, ma anche di restituire dignità al Paese. La tassazione è uno dei fondamenti del patto di cittadinanza e la certezza di quell'obbligo per tutti, non solo per i lavoratori a busta paga, è il primo intervento di equità. Possiamo qui cogliere uno dei tratti che caratterizzano il complesso della finanziaria: restituire dignità allo Stato e alla Repubblica, non solo assicurando che i doveri siano assolti da tutti, ma anche garantendo la qualità dell'azione pubblica. Si è tanto discusso della reintroduzione della riforma Bassanini sull'organizzazione del Governo e in troppi si sono fermati alla superficie dell'intervento, cioè alla riduzione del numero dei Ministri. Vorremmo, invece, sottolineare come quella scelta, se sarà rispettata non solo dal prossimo Governo, ma dai Governi che negli anni si succederanno, darà un forte impulso alla qualità dell'opera e dell'azione dell'amministrazione. Il punto non è il numero, ma la stabilità. Ancora oggi il processo di separazione tra i Ministeri è in corso e così è stato per il Governo precedente e per quello prima ora. Anni persi a spostare uffici, personale, carte. Il punto qualificante non è ridurre il numero, ma assicurare che qualunque Governo sarà alla guida del Paese si troverà a gestire una macchina efficiente, stabile nel tempo, i cui meccanismi sono solidi. Insieme al principio di separazione dei poteri, due poli compongono lo Stato democratico: da un lato la volontà del popolo, che si esprime attraverso gli organi politici, dall'altro un'amministrazione terza, che non segua interessi particolari. È la lezione di altri Paesi, come per esempio la Francia, dove l'intangibilità dell'amministrazione si accompagna ad una chiara distinzione dei ruoli. Così come la scelta, da un lato, di stabilizzare chi oggi opera nell'amministrazione in modo precario e, dall'altro, di assumere, da oggi, solo a tempo indeterminato non è solo una scelta importante sotto il profilo sociale, ma anche dal punto di vista della qualità dell'amministrazione. Il nodo della precarizzazione delle vite e del futuro di intere generazioni si para di fronte a noi con forza e non dare risposte efficaci sarebbe non solo segno dell'inadeguatezza della politica, ma anche e soprattutto gesto colpevole e irresponsabile nei confronti di alcuni milioni di cittadini oggi incapaci di programmare con Ma non c'è solo questo: un'amministrazione dello Stato che fondasse i propri servizi su personale precario, che oggi c'è e domani chissà, diviene precaria anch'essa e i diritti dei cittadini diventano labili, inesigibili. La battaglia per la stabilizzazione non inficia, ma rafforza l'efficacia dell'amministrazione anche considerato che quei lavoratori stabilizzandi dovranno affrontare, come impone la Costituzione, adeguate prove selettive. Con questa finanziaria si afferma la necessità, allora, di una pubblica amministrazione solida e speriamo anche sobria. Con la riduzione delle indennità dei consiglieri comunali e l'eliminazione dei contributi a carico delle amministrazioni locali da un lato, e con il tetto agli stipendi dei *manager*, dall'altro, si riconducono a buon senso, in modo non demagogico, gli effetti perversi di un certo federalismo della spesa che ha minato gravemente la credibilità della politica. Così, a livello centrale, anche il punto di equilibrio saggiamente raggiunto sui fondi di dotazione per gli organi costituzionali che si sono impegnati ad una riduzione della proprie spese è un messaggio importante, ottenuto senza metterne in discussione l'autonomia, che deve essere gelosamente preservata. Risorse dall'evasione fiscale, un impegno per garantire diritti e assicurare che ciascuno si faccia carico dei doveri, un'amministrazione più efficiente, una gestione della cosa pubblica più sobria: queste sono le premesse che abbiamo posto per una politica seria e non demagogica. È con questo patrimonio di autorevolezza che si possono costruire politiche di redistribuzione e impegni per il futuro che diano risposte concrete alle domande del Paese.

che incide in modo indifferenziato rispetto al reddito e alle condizioni di patologia dei cittadini. Sgombrare il campo da questo strumento significa riaffermare il diritto universale alla salute, uno dei fondamenti del nostro sistema di *welfare*, che non vogliamo smantellare, ma anzi rafforzare con decisione. Il secondo è quello per la casa: riduzione dell'ICI e detraibilità degli affitti, insieme al piano di edilizia pubblica deciso nel decreto fiscale, disegnano un intervento complessivo rispetto a quella che è oggi una delle più gravi emergenze sociali. Oggi una casa pesa tremendamente sui redditi dei cittadini. Secondo il Sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari (SUNIA), per pagare l'affitto di casa se ne va più della metà dello stipendio, e si sfiora l'80 per cento dell'intero reddito di una famiglia operaia per affittare nella periferia delle grandi città; per l'acquisto, dal 1970 al 2003, il valore assoluto dello stesso appartamento è cresciuto di 35 volte. Dietro questi numeri ci sono drammi familiari, difficoltà nel selezionare cosa sia prioritario nella spese di casa, privazione di molti beni, spesso anche di quelli primari. Oggi invertiamo la tendenza, con un intervento generalizzato che dà nuovamente fiato alle famiglie e ai cittadini. Un terzo intervento è rappresentato dall'impegno ad investire il gettito supplementare, frutto della lotta contro l'evasione, nella riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente. Come nella legge finanziaria 2006 avevamo deciso di destinare l'extragettito alla riduzione fiscale generalizzata (e oggi ottemperiamo a quell'impegno attraverso gli interventi sulla casa), così ora guardiamo in faccia ad uno dei problemi più drammatici del nostro tempo, cioè la contrazione del potere d'acquisto dei redditi da salario, come fonti inaspettate, ma di grande saggezza e autorevolezza, ci hanno ricordato pochi giorni fa. In una riedizione di antiche politiche dei due tempi, le imprese, tra questa e la precedente finanziaria, hanno ricevuto significative riduzioni fiscali. Ora affermiamo con nettezza che inizia il secondo tempo, quello della restituzione a chi, con il proprio lavoro e la propria fatica, costruisce quotidianamente la ricchezza del nostro Paese. L'altra faccia di questa medaglia sarà la prossima tornata contrattuale, che deve essere caratterizzata da un maggiore equilibrio tra il reddito di chi lavora e i profitti di chi investe. Infine, nell'ampio intervento rappresentato da questa finanziaria, rischia di essere messa in disparte la questione del sistema della conoscenza e della cultura, unica strada che indica al Paese un futuro. Con più di un miliardo e mezzo in tre anni destinati all'Università si inverte una tragica tendenza iniziata dalla precedente amministrazione di ritenere il sapere un costo e non un investimento. Oggi diamo un messaggio di segno opposto. Dall'altro lato, con gli interventi a favore del cinema e della cultura riaffermiamo quel legame costitutivo della comunità nazionale che è stato ed è il nostro patrimonio di idee e opere. Serietà, autorevolezza, sobrietà: questi sono i valori che noi troviamo nel disegno di legge finanziaria e che il passaggio in Commissione bilancio prima e ora in Aula non offusca, ma conferma. Ora, con questo dibattito, affermiamo di fronte al Paese il valore di una politica che, senza demagogia, risolve i problemi e dà risposte a bisogni e ad

signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge finanziaria per il 2008, che stiamo qui discutendo, contiene certamente alcuni punti interessanti e importanti per lo sviluppo del Paese. Si tratta di punti importanti per un Paese che si vuole moderno, attento agli impegni di stabilità finanziaria assunti in sede europea desideroso di concretizzare il principio di uguaglianza e di equità sociale che sta alla base della nostra Carta costituzionale. Condivisibili sono alcune linee tracciate dalla prossima finanziaria: responsabilizzazione della politica e dei cittadini, riduzione dei divari che minano ancora la nostra società e il nostro territorio, riduzione della pressione fiscale, razionalizzazione della spesa pubblica, rilancio delle imprese e dell'economia, attenzione ai giovani, alle fasce sociali più deboli e alle famiglie. Non è un risultato perfetto che soddisfi appieno ciascuno di noi o tutte le componenti del Paese indistintamente e contemporaneamente. Chi governa ha il dovere di ascoltare, di valutare i diversi interessi, di mediare per giungere a soluzioni eque e possibilmente condivise. In questo, nel metodo, bisogna dare atto al Governo di avere voluto e saputo ascoltare. Al Presidente della Commissione bilancio e al relatore va riconosciuto il merito di aver organizzato bene i lavori, permettendo la conclusione dell'*iter* previsto in Commissione. Ciò ha permesso di giungere ad un disegno di legge che ritengo essere significativamente migliorato

massimo 12 Ministri e 60 componenti. È un segnale forte e da non ignorare che vuole concorrere alle esigenze di ridurre i costi della politica. È un sacrificio reale ed apprezzabile per chi conosce le responsabilità e gli impegni concreti che quotidianamente incombono sulle persone che assumono il ruolo di Governo e di amministrazione. L'energia e l'ambiente sono le grandi sfide del nostro tempo e la finanziaria le raccoglie intervenendo attraverso misure mirate, definendo linee generali e azioni specifiche.

La famiglia, nucleo basico della nostra società, e la realizzazione civica di ogni singolo cittadino possono trovare un nuovo slancio nelle politiche in favore di asili nido e di assistenza all'infanzia, nelle iniziative volte ad assicurare l'accesso alla casa e in quelle a favore dei giovani. Il Governo dovrà assicurare successivi impegni già delineati da specifici ordini del giorno in merito a questi temi. l'esenzione dal pagamento dei *ticket* sanitari e fondi per affrontare le patologie dei lavoratori che hanno subito i danni della presenza di amianto. alla politica fiscale, credo sia da valutare con soddisfazione l'avviata inversione di tendenza sulla pressione fiscale. Tutta l'azione condivisa della lotta all'evasione fiscale deve essere assolutamente accompagnata da misure sostanziali di riduzione delle imposte. Sono non soltanto misure giuste nel rispetto del principio di equità, ma anche valide iniziative in grado, insieme con le altre previste dalla finanziaria, di condurre ad una società più coesa e, per questo, con meno tensioni interne e ad una società più sana e dinamica. montagna, delle autonomie, delle minoranze linguistiche e culturali e della situazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ritengo si sarebbe potuto fare di più sia sia per le misure specifiche e puntuali che sono, comunque, previste dal disegno di legge, ma soprattutto in termini di sistema, di mutamento di visione, di maggiore e corretta considerazione di questi quattro elementi che non solo devono essere oggetto di interventi, ma che devono essere considerati attori politici coinvolti e rispettati nel processo di rafforzamento e di coesione del Paese. alla montagna, si rifinanzia il Fondo per la montagna e si riconducono le agevolazioni fiscali per i combustibili da riscaldamento nei Comuni montani e per il teleriscaldamento. Queste misure sono degne di importanza, ma è necessario procedere rapidamente in termini globali sulla materia, come previsto dal disegno di legge n. 1607 del 31 maggio scorso, recante «Misure a favore dei territori di montagna e delega al Governo per l'adozione di un codice della legislazione sulla montagna». I popoli della montagna non vogliono contribuiti, non vogliono essere identificati semplicemente come coloro che vivono in aree disagiate; essi vogliono che sia riconosciuta la loro specificità, la loro autonomia, la loro cultura, che sia ascoltata la loro voce. Ciò che più serve è riconoscere alla montagna la sua diversità, riconoscerle il diritto di sottostare a regole diverse in grado di sviluppare le proprie potenzialità sulla base di linee di governo e di sviluppo create e condivise dagli stessi montanari. Aspettiamo impegni e risposte concrete da parte del Governo su questi temi. Vengo ora alla riforma delle Comunità montane, introdotta nel provvedimento quale contributo alla riduzione dei costi della politica. Trattandosi di una riforma di carattere ordinamentale sarebbe stato molto più opportuno trattare questo tema in sede più appropriata. È necessario riorganizzare le Comunità montane tenendo in considerazione alcuni princìpi fondamentali: salvaguardare e valorizzare il ruolo e le competenze regionali in materia, indicare dei criteri generali di indirizzo affinché le Regioni definiscano in modo articolato il territorio montano, garantire il sistema montagna, che è risorsa del Paese, condizione che la montagna sia viva, siano garantiti i servizi essenziali e sia incoraggiata l'attività economica. La montagna non è un parco giochi, né solo una riserva ambientale naturalistica, ma è un territorio dove vivono e operano comunità attive e radicate, che gestiscono un territorio difficile e delicato, ma ricco di risorse e di culture.

affinché le differenze del nostro Paese possano apportare, ognuna, il loro vero contributo positivo allo sviluppo democratico ed economico. Per le autonomie differenziate, quelle storiche, mi permetto di fare un appunto. Una norma di salvaguardia è generale nel riconoscere la forza delle rispettive prerogative. Disposizioni particolari in termini di Patto di stabilità interno ne rispettano l'autonomia e ne fanno una fucina di sperimentazione di nuovi assetti nei rapporti con lo Stato. Interventi in materia di IRAP e di ICI non ignorano la peculiarità della loro autonomia finanziaria, nel senso di maggiore autonomia e maggiore assunzione di responsabilità. punti qualificanti nel risultato, ma un po' meno nel metodo perché, ancora una volta, si è dovuto vigilare ed intervenire affinché il testo della finanziaria non ignorasse le prerogative costituzionali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Non è segno di attenzione politica che a distanza di 60 anni la Repubblica non abbia ancora metabolizzato le autonomie speciali, capito la loro posizione, accettato il messaggio che i Padri costituenti hanno fissato con il loro riconoscimento. Non è segno di maturità politica voler continuare a considerare privilegi quelli che sono diritti: diritti, princìpi costituzionali quelli che concernono la montagna, le autonomie territoriali, le minoranze, le autonomie speciali. Non ignoriamo questo messaggio, non ignoriamo questa necessità che è importante per tutti: per la Repubblica nel suo insieme e per ciascuna di queste sue particolari componenti. In qualità di unico senatore della Regione autonoma Valle d'Aosta, richiedo la stessa attenzione per la mia Regione che assume in sé, da sola, tutte le dimensioni: è montagna, è minoranza, è autonomia, è autonomia speciale. Le agevolazioni per la montagna di cui ho parlato, le regole particolari per il rispetto del Patto di stabilità interno, l'aver riconosciuto la specifica posizione dell'università della Valle d'Aosta e di quella di Bolzano, l'attenzione ai riflessi sulla Valle d'Aosta conseguenti alle nuove politiche fiscali e alle politiche di messa in sicurezza del territorio, l'auspicata realizzazione di importanti opere viarie e ferroviarie (che toccano la Valle d'Aosta, ma che sono di interesse generale per l'intero Paese) sono per me altrettanti punti di soddisfazione, di dimostrazione che il Governo e la maggioranza hanno saputo ascoltare la nostra voce, comprendendo le nostre ragioni. Voce e ragioni delle minoranze linguistiche e culturali, della montagna, delle autonomie speciali, voci che vogliono essere in armonia con il Paese e ragioni che attraverso la salvaguardia delle diversità, mirano a concorrere alla crescita dell'Italia. Non sono ossessionato dalla difesa gratuita delle differenze, quanto piuttosto - questo sì - dal rispetto dei valori costituzionali, dai valori che queste differenze riconoscono e tutelano, valori che hanno provato tutta la loro forza nella vita repubblicana, valori che, se ignorati, non possono avere altro effetto che quello di condurre ad un Paese e ad una società più povere, perché uniformate ad una pretesa ed artificiale eguaglianza. In conclusione, il mio giudizio politico sulla finanziaria è di un moderato ottimismo. Ascolterò con attenzione le repliche del Governo che invito ad assumere impegni per valorizzare il ruolo delle autonomie speciali, un impegno per la montagna in generale, che non reclama privilegi ma la valorizzazione delle sue grandi potenzialità, un impegno a garantire la specificità del nostro sistema Valle d'Aosta nel suo complesso secondo un accordo dai contenuti precisi che va assolutamente rispettato quale condizione per continuare ad assicurare un leale sostegno a questo Governo e a questa maggioranza.

la manovra di bilancio in esame rappresenta l'ennesima occasione perduta dal Governo Prodi per adottare misure in grado di sostenere ed incentivare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. I timidi segnali positivi provenienti dal mondo della produzione sono ancora una volta ignorati, la pressione fiscale rimane su livelli molto alti - il 43 per cento - e non ci sono interventi seri a favore delle famiglie. Sappiamo che ciò è dovuto alla necessità di tenere in piedi questa variegata e litigiosa maggioranza di cui il Governo è ostaggio, situazione che impedisce l'adozione delle riforme necessarie al Paese. L'instabile equilibrio della maggioranza si basa sul compromesso tra le sue diverse anime e lo spazio di manovra del Governo è ristrettissimo, limitandosi all'ordinaria amministrazione, senza alcuna visione strategica. Il risultato è una manovra priva di sostanza, composta da un coacervo di misure frammentarie, di breve respiro, che allontanano il Paese dal percorso di risanamento finanziario e di riduzione del rapporto *deficit*-PIL. Prima di varare la manovra il Ministro dell'economia e delle finanze aveva elaborato il Libro Verde, ponendo quale obiettivo principale la revisione dei criteri di determinazione della spesa pubblica al fine di operare i necessari tagli, la semplificazione della struttura del bilancio con una maggiore attenzione al risultato da conseguire piuttosto che al centro di spesa e la definizione di indicatori quantificabili e soprattutto verificabili *ex post*. Ma alla luce del documento presentato dal Governo possiamo dire che il Libro Verde è rimasto in gran parte lettera morta. E se è vero che la nuova suddivisione in missioni e programmi ne ha reso più semplice la lettura, spostando l'attenzione da chi gestisce le risorse a cosa si fa con le risorse, è anche vero che della *spending review* non vi è traccia. In che cosa consiste la razionalizzazione della spesa pubblica e dove sono i grandi tagli annunciati è difficile dirlo. Al contrario la manovra comporta un aumento della spesa primaria, non vi è traccia di risparmi, se non quelli del tutto ipotetici e fantomatici che dovrebbero derivare dalla gestione degli immobili pubblici. In realtà il Governo rinuncia ad affrontare il nodo della spesa e anzi rinvia il rientro dal disavanzo, unica misura davvero necessaria per creare condizioni favorevoli alla crescita. Infatti, il risanamento dei conti pubblici e la conseguente riduzione del debito è il presupposto essenziale dello sviluppo. Ma la strada intrapresa dal Governo va nella direzione esattamente opposta, con l'adozione di misure di carattere espansivo, dall' effetto per lo più estemporaneo, piuttosto che di compressione della spesa; cosa, questa, che rallenterà la crescita e lo sviluppo. Di questa manovra, quindi, contestiamo la scelta di fondo, tesa a utilizzare l'extragettito per finanziare ulteriori spese piuttosto che per risanare il debito pubblico. I rilievi del presidente della Corte dei conti sono chiari ed inequivocabili al riguardo. Rimandare il rientro dal debito migliorando il rapporto *deficit*-PIL è una scelta di politica economica miope, una rinuncia ad investire nel futuro. Ma, in effetti, a ben guardare nella manovra manca una vera e propria politica . economica, se essa vuol dire adottare scelte strategiche, strutturali e durature per il Paese. Quello che troviamo - sconti fiscali, *bonus* per gli incapienti, sconti sugli affitti - sono interventi a macchia di leopardo, diretti ad accontentare una parte della maggioranza senza scontentarne altre, misure contingenti, una *tantum*, dietro alle quali non c'è un disegno coerente e unitario. Queste misure non aiutano chi ha veramente bisogno: non aiutano le imprese e non aiutano le famiglie. I tagli dell'IRES e dell'IRAP non incentivano la ripresa e la competitività, poiché se da una parte semplificano dal punto di vista burocratico gli adempimenti fiscali a carico delle imprese, dall'altra sono a costo zero, per cui il gettito deve rimanere invariato. Non si introduce, quindi, alcuna riduzione del carico fiscale, perché l'abbassamento dell'aliquota è accompagnato dalla rimodulazione e dall' allargamento della base imponibile, attraverso la riduzione degli oneri deducibili. Si tratterà solo di vedere chi guadagna e chi perde, ovvero quali imprese saranno favorite perché pagheranno di meno (sicuramente, quelle fortemente capitalizzate e che hanno scarsamente investito) e quali quelle svantaggiate che pagheranno di più (ossia, ancora una volta le piccole e medie imprese, che hanno effettuato investimenti o che, peggio ancora, si trovano in difficoltà). Non si aiutano le famiglie, cui non viene prestata la dovuta attenzione. Le misure redistributive a favore degli incapienti e gli sconti fiscali sugli affitti per i giovani sono a carattere temporaneo, e neanche in tal caso si allenta la pressione fiscale. Noi dell'UDC siamo convinti - e lo ripetiamo da tempo - che una politica fiscale equa debba avere come soggetto di riferimento il nucleo familiare, su cui va modulato il prelievo e su cui vanno calcolati i benefici. Per sostenere le tante famiglie italiane oggi in grande difficoltà occorrerebbe tener conto del quoziente familiare, ripensando l'intero sistema fiscale, e non adottare interventi *spot* di dubbia efficacia. Anche il taglio dell'ICI, rispetto al quale è stato eliminato il tetto dei 50.000 euro di reddito, è una misura condivisibile in via di principio, ma non era certo tra le cose urgenti da fare, anche perché incide sull'unica vera entrata propria dei Comuni, e la conseguenza sarà un innalzamento delle imposte locali per compensare la diminuzione conseguente del gettito. In materia energetica non viene previsto nessun intervento rilevante se non la proroga di qualche incentivo che certo non serve a risolvere i problemi seri di approvvigionamento del nostro Paese e di aumento dei costi legati all'energia che richiederebbero ben altre scelte, come il ricorso all'utilizzo del nucleare. Nessuna misura di incentivo allo sviluppo e alla crescita neanche nel campo delle infrastrutture, dove si continuano a effettuare ingenti trasferimenti per ripianare i *deficit* delle grandi aziende. L'esame in Commissione bilancio ha inoltre peggiorato il quadro, poiché la maggioranza, con un comportamento irresponsabile, ha introdotto alcune modifiche che hanno fatto lievitare la spesa. Altro che manovra *light*! È stato stabilizzato un ulteriore numero di precari, sono state previste ulteriori assunzioni della pubblica amministrazione. Molti di questi interventi aggravano l'entità della manovra e su molti di essi si pongono problemi di copertura, su cui spero il Governo ci sappia dare i necessari chiarimenti. Non parliamo, poi, dei tagli ai costi della politica, passati dall'iniziale risparmio di 1,3 miliardi di euro agli irrisori 419 milioni! Di qui all'approvazione definitiva della manovra chissà quante altre spese verranno fuori, visto che il Governo non è in grado di controllare l'assalto alla diligenza in sede parlamentare, costretto a trattare, al limite del ricatto, su ogni singola questione. In conclusione, analizzando questa manovra non si può far altro che constatarne tutta l'inconsistenza, la frammentarietà e le contraddizioni, che poi riflettono lo stato di questa maggioranza. Se la politica di questo Governo si basa sulla speranza di accumulare tesoretti per poi dilapidarli senza alcun reale vantaggio per l'economia, credo che ci sia anche stavolta riuscito, ma proprio per questo c'è da essere davvero preoccupati per il futuro soprattutto, perché il prezzo di queste scelte sbagliate le paga il Paese, che rischia di perdere il treno della timida ripresa in atto, il che ci sembra davvero veramente troppo!

la legge finanziaria pone un freno allo sviluppo del sistema della comunicazione nel nostro Paese e colpisce pesantemente le imprese del comparto radiotelevisivo, in perfetta coerenza con la politica dissennata e punitiva intrapresa con ostinazione sin dall'inizio del suo mandato dal Ministro delle comunicazioni. Le linee guida di questa politica anacronistica sono in discussione in Parlamento con i disegni di legge n. 1825 alla Camera e n. 1588 al Senato sulla riforma RAI (che in realtà riforma ben poco, se non in senso peggiorativo, accentuando ipocritamente la dipendenza del servizio pubblico Tutte le imprese del sistema sono insoddisfatte per le omissioni e per le vessazioni contenute nei diversi provvedimenti, le cui conseguenze saranno assai pesanti e nefaste sul comparto radiotelevisivo del nostro Paese, mortificato e residuale nell'ambito di un mercato sempre più sovranazionale. L'Europa si sta convertendo alla tecnologia televisiva digitale. Ragioni di carattere economico, sanitario, ambientale e sociale concorrono ad una trasformazione oramai ineludibile. Nella precedente legislatura il Governo aveva attuato un'adeguata politica di incentivazione allo sviluppo della nuova tecnologia, in una logica di sistema Paese perfettamente inserito in un contesto internazionale. Questo Governo, al contrario, sembra avere obiettivi opposti. Non prendete alcuna misura per l'effettivo sviluppo della tecnologia digitale terrestre, con il rischio di relegare il nostro Paese in una situazione di assoluta marginalità tecnologica. L'incremento di appena 20 milioni (quindi risibile) del fondo di cui all'articolo 39, comma 2, appare meramente simbolico e del tutto insufficiente ad accelerare lo sviluppo del digitale. A questo si aggiunge lo spostamento dello *switch off* al 2012, previsto dal decreto legge collegato alla finanziaria che abbiamo approvato qualche giorno fa. Uno spostamento per certi versi necessario, che si sarebbe però dovuto accompagnare con un piano progressivo di digitalizzazione, per dare certezze alle imprese televisive, al sistema industriale che costruisce gli apparati e soprattutto a un'utenza sempre più disorientata. Tutte le imprese italiane, senza eccezione, da tempo chiedono che, tale spostamento venga accompagnato da un piano credibile per aree geografiche. L'abbandono dell'analogico per aree geografiche ha già dimostrato di essere un percorso efficace: lo spostamento di "RAI 2" e "Rete 4" a Cagliari e ad Aosta solo in digitale è stato un successo. A marzo 2008 cesseranno le trasmissioni analogiche di tutte le reti in tutta la Sardegna e da ottobre in tutta la Valle d'Aosta. Altre Regioni e Province autonome hanno dichiarato il loro interesse al passaggio al solo digitale entro il 2009. Lo spegnimento dell'analogico per aree geografiche cadenzato da qui al 2012 è l'unico strumento realmente efficace per consentire all'Italia di condividere il processo europeo di progressivo abbandono della vecchia TV analogica. La pubblicazione del Piano di spegnimento consentirebbe anche un efficace riordino delle frequenze e un dividendo per utilizzi ulteriori rispetto alla conversione delle reti televisive attualmente operanti, ma darebbe soprattutto un quadro di garanzia a tutti gli operatori. Senza date intermedie sicure e piani coordinati con strumenti attuativi, lo spostamento al 2012 resta solo un ennesimo e poco credibile rinvio. Nessuna ragione logica può giustificare un simile atteggiamento. In realtà, sembra che qualche *pasdaran* favorevole alla distribuzione gratuita di frequenze analogiche agli amici degli amici, cosa spudoratamente contenuta nell'orribile disegno di legge Gentiloni giacente alla Camera, ritenga che un processo di digitalizzazione progressivo possa impedire da subito la liberazione delle frequenze, da offrire in gentile omaggio alle organiche e allineate "Europa 7" e "Rete A", tanto per non fare nomi. Del tutto trascurato è poi il settore rappresentato dalle emittenti radiotelevisive locali. Ai 10 milioni di aumento del finanziamento della legge n. 448 del 1998 previsto dalla legge finanziaria non si sono però accompagnate quelle ben più importanti norme di snellimento delle procedure che Alleanza Nazionale aveva chiesto per consentire l'erogazione effettiva dei pagamenti dei contributi alle emittenti. Per l'incapacità del Ministero a fornire nei tempi pareri e direttive applicative, le emittenti non hanno ancora ricevuto un solo euro delle somme di loro spettanza per l'anno 2006; un ritardo record, inammissibile e fortemente penalizzante per le imprese, le cui responsabilità sono da attribuire *in toto* ad una gestione a dir poco approssimativa del Ministero. Alle carenze e alle dimenticanze più o meno volute si accompagnano poi una serie di norme demagogiche e anticostituzionali, che incidono sulla libertà di iniziativa e di investimento delle imprese, a beneficio di quella parte della cinematografia nazionale che, refrattaria alla logica del mercato e della concorrenza, vuole non solo la facile assistenza diretta dallo Stato, ma anche quella indiretta, attraverso l'imposizione di pesanti obblighi da far gravare sulle imprese televisive, considerate come vere e proprie galline dalle uova d'oro cui attingere a piacimento. Le norme che prevedono un rafforzamento degli obblighi di investimento e di programmazione delle imprese televisive nelle opere di produzione europea e italiana, previste dall'articolo 40, oltre che estranee alla materia, sono il frutto della mentalità dirigistica tipica di questo Governo. Accanto a produzioni di indubbio valore qualitativo e di mercato, purtroppo nella cinematografia italiana vi è anche una forte componente di soggetti che non riesce a liberarsi dalla logica dell'assistenzialismo. Non è certo con il vincolo di programmare in percentuale obbligata i film italiani in *prime time* che si aiutano i cittadini e il cinema. Se meritevoli, tali produzioni andranno comunque negli orari di buon ascolto; altrimenti no. La portata di tali disposizioni andrebbe pertanto rivista per attenuarne, anche a livello operativo, gli onerosi impegni gravanti sulle emittenti in una logica di ragionevolezza. Le proposte di Alleanza Nazionale vanno in questo senso, ma la maggioranza e il Governo sembrano ostili. L'imposizione di ulteriori misure stringenti e coercitive nei confronti delle imprese televisive le costringerebbe ad atteggiamenti oltremodo difensivi e di fatto ostativi verso un prodotto come l'opera cinematografica. Va inoltre considerato che la discriminante in favore delle opere cinematografiche concepite nella logica della sola distribuzione in sala è fuorviante. Tutta la produzione audiovisiva infatti, al di là del suo utilizzo iniziale e finale, vede come protagonisti gli stessi soggetti (autori, sceneggiatori, attori e produttori) e non si comprendono le ragioni per cui il prodotto non concepito originariamente per la sala non debba avere la stessa dignità dell'opera cinematografica propriamente detta. Tra l'altro, esistono e potranno esistere film diffusi sia nelle sale che in televisione. Ai fini dell'obbligo di investimento e di programmazione non può quindi essere considerata come discriminante la sola uscita nelle sale. La RAI è ovviamente colpita da questa legge finanziaria; peraltro, all'ultimo momento, con un emendamento approvato in Commissione, è stato fissato un tetto di 274.000 euro ai compensi per i dipendenti e i consulenti. Contro tale norma c'è stata una levata di scudi del direttore generale, Claudio Cappon, in un'intervista su «la Repubblica». In ogni caso se la RAI ritiene di doversi considerare un'azienda commerciale come le altre, quindi di liberalizzare i compensi per i propri consulenti, dovrebbe anche pensare di rinunciare al canone. affermando che nulla è previsto all'interno di questa finanziaria per combattere il fenomeno dell'evasione del canone.

Signor Presidente, per brevità concentrerò il mio intervento su un solo tema, sul quale del resto non è la prima volta che mi intrattengo: la montagna. Lo faccio volentieri, in quanto abbiamo l'occasione, non frequente, di avere come ascoltatrice direttamente la responsabile della delega per la montagna, la ministra Lanzillotta. Debbo dire, Ministro, come uomo che s'interessa di montagna da molto tempo, prima al Parlamento europeo e ora al Parlamento italiano, che profondamente deluso per il disinteresse o - diciamolo in termini più eleganti - la scarsa attenzione che questo Governo in un anno e mezzo di attività ha destinato a tutte le risorse e tutte le attività che riguardavano la montagna. disinteresse si è poi concretizzato anche in questa finanziaria in alcuni interventi a dir poco inopportuni, come anche alcuni colleghi della maggioranza hanno osservato. Ciò è ancora più strano e amareggia in misura maggiore in quanto perfino l'Unione Europea, che si era distinta in passato per una totale indifferenza verso la specificità della montagna, sta tornando sui suoi passi. L'Unione Europea approvato nel 1998 una risoluzione globale sulla montagna, nel 2001 un'altra risoluzione sull'agricoltura di montagna e, con intervalli sempre più frequenti, torna ad interessarsi di questa specificità; anche perché tra i 10 nuovi Paesi, 12 con i Paesi entrati dal 2004 al 2007, molti hanno caratteristiche di montagna. Non si doveva però aspettare questo evento, in quanto già l'Europa aveva una forte presenza di zone di aree di montagna; il 35 per cento del territorio europeo è considerato di montagna e vi abitano milioni di persone e di cittadini, pari al cento del totale. Va detto che l'Europa ha fatto una cosa importante inserendo la specificità della montagna prima nella Carta costituzionale accanto a quella delle isole ed ora anche nel trattato di della Costituzione da tutti sognata (è una copia sbiadita). In ogni caso, conserva la segnalazione della montagna tra i territori degni di una legislazione particolare; riconosce la specificità e poi ogni Paese membro fa la sua parte. L'Italia, fra i Paesi di montagna, sicuramente non ha nulla da invidiare a nessuno, visto che il del suo territorio è considerato di montagna; vi abitano ben 12 milioni di cittadini, pari al 18 per cento del totale nazionale; produce, la montagna, il 16 del prodotto interno lordo nazionale; in montagna sono allocate, signora Ministro, il 20 per cento delle aziende agricole italiane, il 35 per cento delle aziende artigiane, cento delle aziende industriali, il 66 per cento delle imprese di servizi e naturalmente c'è il turismo che la fa da padrone, con l'11,8 per cento del fatturato turistico nazionale, grazie a 35 milioni di presenze annue di turisti. La montagna, quindi, non è quell'area depressa che tende la mano che molti vogliono dipingere. La montagna è un sistema sociale ed economico completo e complesso, capace di essere autosufficiente. Ha bisogno di una sola cosa: di qualcuno - e il Governo è titolato a farlo - attraverso le Regioni che crei la famosa rete di connessione, di collegamento tra tutti i settori che si occupano di montagna. Ecco quindi che non siamo qui a pietire - l'hanno detto anche colleghi della maggioranza - nulla in più di quello che spetta ad altri territori, ma certamente un riconoscimento esplicito, chiaro della specificità della montagna. Purtroppo questa finanziaria non testimonia, non documenta questa intenzione. Partire adesso dall'articolo 13, che riguarda la riforma, così definita, delle Comunità montane, è fin troppo facile. Che in questo campo vi fosse bisogno di interventi di riordino, di ridimensionamento siamo tutti d'accordo. Ma partire con una riforma inserita in una finanziaria è come prevedere la riparazione di un rubinetto nel complesso di ristrutturazione di un grattacielo. Chiaramente sfugge e non potrà essere mai una riforma oculata e precisa. Noi siamo ancora favorevoli, se è possibile recuperare un emendamento *ad hoc*, signor relatore, allo stralcio totale dell'articolo 13 e non per dare un segnale di critica verso il Governo, anche se dal mio punto di vista tutte le critiche sono plausibili, ma per consegnare questa delicata e complessa materia ad un disegno di legge organico - disegno di legge che è stato già depositato in Senato di cui il primo firmatario è il

Inoltre, molti hanno già osservato che la finanziaria è una legge di carattere amministrativo, che non può inserire elementi e contenuti di carattere ordinamentale. Quindi, si corre anche il pericolo che, subito dopo l'approvazione della finanziaria, con queste proposte le Regioni - l'hanno già preannunciato in maniera esplicita - intervengano con ricorsi alla Corte costituzionale. Perché allora andare incontro ad un episodio così sgradevole con una iniziativa legislativa che scontenta alla fine tutti? Perfino il Servizio di bilancio del Senato ha osservato che taluni passaggi, soprattutto quelli amministrativi, abbisognano di norme apposite approvate dalle Regioni. dobbiamo lasciar perdere in questa finanziaria il tema montagna e Comunità montane, per consegnarlo o alla legge sulla montagna o ad una occasione ulteriore, come la legge già depositata e incardinata sulla riforma dei piccoli Comuni, insomma in un contesto nel quale con maggiore competenza e serenità si possono affrontare detti problemi. E poi eliminiamo tutto quello che non è montagna, quello che rappresenta oggi una aneddotica fin troppo noiosa tanto viene sfruttata, come i Comuni di Sperlonga, Porto Santo Stefano, l'isola d'Elba, Palagiano. È vero: tagliamo i Comuni costieri, non sono più di montagna. Ma non possiamo - come come si usa dire in questi casi con una allegoria fin troppo abusata - buttare il bambino con l'acqua sporca: via tutte le Comunità montane, così siamo sicuri di colpire anche quelle che non meritano tale etichetta. C'è poi l'aspetto finanziario, signora Ministro, che non trova d'accordo il Governo e l'UNCEM, un organismo che - ci perdoni - per noi è ancora un punto di riferimento molto importante e attendibile. Noi viviamo in montagna e siamo abituati a ragionare con questo organismo sovracomunale, reputandolo un riferimento serio.

come consigliere comunale esclude quella della Comunità montana. Questa è la grande differenza di filosofia tra Governo e UNCEM e anche tra noi. Per quanto riguarda l'abolizione di queste Comunità montane,

per non avallare le mie crude dichiarazioni di un vostro disinteresse totale verso la montagna. Signor Presidente, la prima proposta è di aumentare la dotazione del Fondo nazionale della montagna, decisamente esigua, soprattutto per quanto riguarda gli anni futuri.

per avallare la vostra affermazione di voler valorizzare la ricerca, tanto più che questa è una ricerca mirata sulle problematiche della montagna. Perché, poi, al CAI (Club Alpino Italiano),

ha trovato le risorse per modificare, intervenire sulle condizioni di vita di questi cittadini del nostro Paese

si aspetta non in forma passiva, ma attivamente, lottando quotidianamente nelle condizioni in cui si trova. Credo che questo debba essere l'asse della politica di questo Governo di qui in avanti. Pur tuttavia, nella finanziaria ci sono alcuni segnali blandi, frammentari, ma importanti, perché sembrano andare nella direzione di un ascolto, di una risposta a chi produce la ricchezza del Paese, a chi produce la stabilità del Paese, ma non si vede riconosciuto alcunché. In questa finanziaria è mancata la tassazione della rendita ai livelli europei: con questa avremmo potuta finanziarie

agli incapienti; è una restituzione dovuta nella misura in cui altrimenti lo Stato, attraverso la fiscalità, non sarebbe stato in grado di ridare loro quello che per loro condizione non possono ottenere, ma non ha nemmeno restituito il *fiscal drag*, cioè un prelievo ulteriore, forzoso, sul reddito delle persone a lavoro dipendente. Purtroppo - ne discuteremo più avanti - non ci sono provvedimenti seri sugli ammortizzatori sociali e sulla flessibilità del lavoro. Mi pare che questi siano gli elementi di maggiore insicurezza

proponevamo una copertura che riteniamo importante venga discussa, per la quale l'INPS, che ha un fondo per la maternità, lo usi esattamente per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Non posso quindi che dolermi e chiedere che venga accolto perlomeno l'ordine del giorno che presenteremo sui congedi parentali, sperando così che sia alla Camera, sia nel futuro, questo Governo riesca a lavorare concretamente per migliorare anche la condizione delle lavoratrici.

ho ascoltato con attenzione la breve intervista rilasciata dal ministro Padoa-Schioppa al TG1 delle ore 20 e ho memorizzato una affermazione che egli ha fatto quando, riferendosi al Governo della passata legislatura,

l'infondatezza di questa affermazione e in secondo luogo l'incoerenza del ministro Padoa-Schioppa, che a parole si sforza di apparire un rigorista, mentre nei fatti (contribuendo, come ha contribuito, alle scelte compiute in questi 17 mesi di Governo Prodi) ha avallato una politica dissennata, che ha determinato - ripeto, nei fatti - un aumento della spesa pubblica e della pressione fiscale ed un peggioramento del *deficit*. Andiamo con ordine, signor Ministro. Appena insediato, il Governo Prodi si è molto speso nel denunciare una condizione di sfascio nei conti pubblici, arrivando a fare del vero e proprio allarmismo. Il massimo della denuncia

la loro forza è irresistibile; e, invero, i fatti hanno smentito le sue improvvide dichiarazioni. I conti pubblici ereditati dal Governo Berlusconi non si presentavano come li aveva descritti il Ministro dell'economia, tant'è che le entrate nel 2006 sono state maggiori del 21 per cento delle vostre previsioni, tali da non giustificare una manovra correttiva come quella varata

attraverso tagli alle spese strutturali nei settori strategici (il ministro Padoa-Schioppa ha detto: punteremo a tagliare la sanità, le pensioni, il pubblico impiego, la finanza degli enti locali); a fine settembre il Governo invece ha presentato una finanziaria di 33,4 miliardi di euro, senza tagli alle spese ma con tanti nuovi balzelli, una manovra tutta imperniata sull'aumento della pressione fiscale; a fine ottobre 2006 l'ufficio

È ormai chiaro a tutti, quindi, che la stima del disavanzo 2006 e quella del tendenziale 2007 è stata fortemente inficiata da una sottovalutazione delle entrate.

manovra esagerata per il 2007. Nel corso del 2007, poi, la sottovalutazione delle entrate è diventata talmente evidente che siete stati costretti a rivedere la stima delle entrate di 18,3 miliardi di euro, il cosiddetto tesoretto. Di questo importo, disattendendo purtroppo quanto scritto nella finanziaria dell'anno precedente, grazie anche all'impegno del presidente della Commissione bilancio Morando, anziché destinare le intere maggiori risorse alla riduzione del debito, ne avete finalizzate 13,7 per alimentare la spesa pubblica. Nonostante tutto questo, la rilevante manovra di aumento delle entrate non ha sortito progressi significativi, tant'é che il disavanzo dal 2,5

ha prodotto un forte rallentamento dell'economia reale, certamente più accentuato di quanto si sforza di rappresentare l'ISTAT con i suoi dati ufficiali. Perché

Mi chiedo: è possibile risanare la finanza pubblica e gettare le basi per uno sviluppo aumentando consistentemente le tasse? Certamente no. Non vi è nessun economista di rango che possa proporre una simile ricetta. Purtroppo questa, signor Presidente, è l'impostazione che da sempre la sinistra cavalca, un'impostazione seguita anche da questo Governo, che ci porterà a commettere gli stessi errori commessi all'inizio degli anni '90 anni '90 allorché si tentò di riequilibrare i conti pubblici con un forte inasprimento della pressione fiscale: e il risultato fu - ricordiamoci il 1993 - di produrre deflazione, disoccupazione e ritardare l'ammodernamento dell'apparato produttivo del nostro Paese. Il Governo Prodi sta facendo questo, anzi peggio, perché, avendo sbagliato nel 2006, ha ribaltato l'errore facendo una manovra esagerata a fine dello stesso 2006; nel 2007 ha utilizzato il "tesoretto" per aumentare la spesa pubblica,

la spesa pubblica è aumentata; la pressione fiscale, di conseguenza, è aumentata; il ciclo economico, che nel 2006 dava segni di ripresa, è rallentato al punto che oggi alcuni economisti avveduti cominciano a parlare di inizio di recessione. È propaganda tutto questo, signor Presidente? Non credo. Non credo. Basta leggere con attenzione quanto contenuto nella tabella 3 a pagina 6 della Nota di aggiornamento al DPEF relativo alla manovra finanziaria che voi avete consegnato all'attenzione di questo Parlamento.

di 3,2 miliardi quello del mese di ottobre. Quindi le cose non vanno proprio per nulla bene. Per questi motivi contestiamo questa finanziaria, che non è, come dice il Ministro dell'economia, una finanziaria leggera, bensì una finanziaria falsa e preelettorale.

Per tali ragioni, credo che questa finanziaria forse salverà il Governo per "l'abilità" del presidente Prodi di tenere assieme questa maggioranza così divisa e composita, ma non salverà il nostro Paese.

a criticarla, immaginando di essere in perfetta sintonia con quella parte viva del Paese che produce, che fatica, che si ingegna e che ha sempre meno fiducia nell'operato di questo Governo e di questa maggioranza.

in un'Aula praticamente deserta, che io considero sempre più, da neosenatore, pregna di retorica, ipocrisia e demagogia,

Veniamo a questo tentativo di confronto con il Governo. Come senatore dell'opposizione mi rivolgo al sottosegretario Sartor, innanzi tutto trasmettendogli solidarietà perché è presente dall'inizio della discussione

Poiché già altri hanno parlato di quella relativa alle persone fisiche, ai lavoratori, ai dipendenti delle aziende, da imprenditore permettetemi di soffermarmi sul problema dell'imposizione fiscale alle imprese. Innanzitutto, rilevo

invece in Italia le aliquote fiscali si applicano su una base imponibile che non ha se non

perché il regime di calcolo delle imposte, sia per l'IRES che per l'IRAP, è abbastanza complicato. Mi divertirei a porre ai presenti

tanti anni del calcolo di tali imposte. Per molte imprese, soprattutto per quelle ad alto tasso occupazionale,

in linea con il Governo attuale. Mi riferisco all'associazione delle piccole imprese che nell'Emilia-Romagna ha condotto un'indagine dalla quale è emerso che l'8 per cento delle aziende esaminate, pur presentando bilanci con un utile civilistico rilevante, a seguito dell'imposizione fiscale dichiarano perdite di bilancio. Questo è un argomento caro anche alla senatrice rappresentante degli altoatesini, ma non la vedo in Aula. Spero si informerà su queste cose.

su questa finanziaria e il confronto con il Governo non avviene nel dibattito in Aula. Questo è un Governo sottoposto a un regime di estorsione continua da parte di molti senatori della maggioranza che in questo momento stanno trattando con Padoa-Schioppa queste loro estorsioni per ottenere quello che poi garantirà il voto favorevole al provvedimento. È drammatica questa considerazione, ma è vera perché abbiamo già visto, perfino in Aula, i tentativi di qualche senatore eletto all'estero di ricattare il Governo, così come fanno alcuni altri senatori dissenzienti. Questo non è un Paese civile

Noi abbiamo presentato tre emendamenti: uno relativo all'IRES, uno all'IRAP e uno agli oneri finanziari. Diciamo un'altra cosa: in queste procedure macchinose di elaborazione dei dati ai fini del calcolo delle imposte, questi due, a mio avviso, criminali dell'economia - mi riferisco a Prodi e Padoa-Schioppa che non sono economisti, ma criminali dell'economia per le piccole e medie imprese hanno introdotto delle novità, dimenticando che la piccola e media industria italiana, che è l'ossatura industriale del Paese, è indebitata con il sistema bancario. Ebbene, si sono inventati, tra le altre cose, la possibilità di scaricare gli interessi bancari solo parzialmente: il 30 per cento rispetto al margine operativo lordo

ha un peso degli interessi, visti anche i mercati finanziari, pressoché identico se non peggiorativo. Questi meccanismi che vi inventate servono unicamente a fregare le imprese; siate un po' onesti e cercate un attimo di rivederli perché voi state facendo correre un rischio al sistema industriale italiano. Ci sono alcuni che stanno stimando in circa un milione le piccole e medie imprese che, se venisse approvata questa famigerata finanziaria 2008, chiuderanno i battenti. Siete irresponsabili, se non vi ponete con urgenza questo problema perché poi sapete benissimo Sartor, controlli al suo Ministero - che tutte le pubbliche amministrazioni sono in ritardo con i pagamenti, non rispettano i capitolati di appalto. Stato, pertanto, è inadempiente, le Regioni sono inadempienti, i Comuni sono inadempienti, le amministrazioni provinciali sono inadempienti. Di conseguenza, per la mancanza di liquidità anche tanta impresa italiana è inadempiente con l'altra impresa. Ritroviamo, dunque, condizioni di crisi di tantissime aziende che, con questo meccanismo di calcolo delle imposte, dichiareranno tutte tutte - almeno questo milione stimato - perdite di esercizio, dopo aver chiuso l'utile civilistico con un risultato estremamente positivo.

alta), ponetevi questo problema, sia per l'IRES che per l'IRAP. Gli emendamenti a cui ho fatto riferimento, che sono stati respinti in Commissione, erano finalizzati a mettere un sistema di controllo al calcolo di queste imposte.

al 27,5 per cento deve essere reale e concreta; non dovete falsare i numeri, non dovete cambiare le regole per cui, un po' come per la riduzione dell'ICI, poi si rivedono le tabelle degli estimi catastali e la gente paga più ICI di prima. Gli italiani non sono stupidi, voi potete resistere in quest'Aula ancora per tutto il tempo in cui riuscirete, con le estorsioni che subite dagli stessi senatori della maggioranza,

Come è emerso dalla analisi compiuta dai nostri uffici economici, si tratta di un provvedimento che parte da un presupposto generalizzato - e dunque, sbagliato - che avrà come conseguenza l'ulteriore divaricazione tra Nord e Sud, tra economie forti e economie in fase di ripresa. Il presupposto sbagliato di un provvedimento che alla lunga si dimostrerà iniquo è che la capitalizzazione delle imprese (e quindi la loro solidità) sia omogenea su tutto il territorio nazionale. Con ogni evidenza, si tratta di una filosofia, di un'astrazione, di un'immaginazione, assai lontana dalle condizioni del Paese reale. La situazione vera delle imprese del Mezzogiorno è di una faticosa ripresa quando ancora non sia un'estenuata stagnazione - fondata sull'indebitamento, su condizioni finanziarie difficilissime, su una relazione con il credito, e sopratutto con il credito bancario, che lascia le nostre aziende ai limiti della sopravvivenza. Tutto ciò viene disatteso da un provvedimento fondato sul principio della penalizzazione delle imprese indebitate. Ci si chiede come sia possibile che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia formulato un'ipotesi di lavoro così distante dalla situazione reale. Questo nuovo principio di tassazione non solo avrà come esito la chiusura del Sud che lavora, ma aumenterà in modo scandaloso la già ampia forbice che separa

che sia necessaria una revisione immediata, complessiva e radicale dell'articolo 3 della legge finanziaria in corso di dibattito parlamentare. Naturalmente, non mancherò di far sentire questo grido di allarme ovunque sia possibile dare un contributo concreto che vada dal Paese reale alle sedi istituzionali». La lettera è firmata dall'onorevole Angelo Villani, presidente della Provincia di Salerno, noto esponente di questa novità della politica italiana che è il Partito democratico. Vergognatevi!

Egregio Presidente, colleghi senatori, la legge finanziaria in discussione, così come impostata dal Governo, rappresenta un'autentica delusione per tutti i cittadini italiani, ma soprattutto e segnatamente per quelli meridionali meridionali per i lavoratori dipendenti, per le famiglie e per le imprese. Non mi dilungherò molto nel mio intervento, ma ritengo decisamente necessario marcare alcuni aspetti la cui portata negativa è sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco ai precari e alle misure contenute nella legge: c'è il rischio concreto di creare ulteriori sperequazioni per i lavoratori già svantaggiati. Infatti, la richiesta di aumentare, tramite l'innalzamento dell'aliquota contributiva, il costo del lavoro parasubordinato per scoraggiarne l'uso improprio, non è stata accompagnata, nella finanziaria, da criteri precisi per definire i compensi dei collaboratori. In questo modo l'aumento dell'aliquota verrà scaricato ancora una volta sui lavoratori parasubordinati diminuendo così il loro già esiguo compenso netto. Saranno purtroppo ancora una volta i lavoratori a pagare. Infatti, non c'è alcuna norma volta a stabilire che i compensi dei parasubordinati non siano inferiori a quelli previsti nei contratti collettivi nazionali per i dipendenti che fanno riferimento ad analoghe professionalità. Per le partite IVA individuali, l'aumento sarà ancora più pesante, non essendoci alcun riequilibrio fra quanto pagato dal lavoratore e quanto dal datore di lavoro. Questi lavoratori, a differenza degli altri, dovranno pagarsi per intero i contributi. L'assenza di costi previdenziali a carico dei committenti è quindi un incentivo all'utilizzo improprio di lavoratori con partita IVA individuale. L'aumento della contribuzione non è poi accompagnato da un incremento delle tutele e delle prestazioni sociali a favore dei collaboratori che, a causa delle loro condizioni lavorative, ne avrebbero tratto reale vantaggio. Rimangono pertanto insolute le questioni riguardanti la tutela della gravidanza a rischio per le collaboratrici e il riconoscimento della disoccupazione con requisiti ridotti a lavoratori che si caratterizzano per una forte discontinuità lavorativa.

Nel frattempo però altre critiche arrivano dall'interno del Paese, ma anche da ampi e significativi settori dello Stato. La Corte dei conti critica la scelta del Governo nella manovra 2008 di «rinviare l'individuazione delle risorse necessarie per la definizione dei rinnovi contrattuali del biennio di competenza 2008-2009». Questa scelta, ha detto il presidente della Corte Tullio Lazzaro durante un'audizione sulla finanziaria nelle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato, è «non priva di implicazioni negative rilevanti». Anche per la magistratura contabile per la magistratura contabile non tutto il "tesoretto" può essere dato per scontato. L'avvertimento arriva dalla Corte dei conti, secondo cui ben 3,6 miliardi sui complessivi 5,9 miliardi di extragettito stimati nella Nota di aggiornamento sono a rischio. È stato chiesto al Governo di spiegare se il maggiore incasso sia stato calcolato «tenendo conto dell'andamento di tutte le entrate correnti o dell'aggregato che comprende solo le entrate tributarie e i contributi sociali». Si tratta, ha affermato, di «un dubbio che va chiarito perché in base al monitoraggio condotto dalla Corte dei conti risulta un andamento fortemente negativo delle entrate erariali extratributarie» che nei primi nove mesi del 2007 hanno segnato un calo superiore al 23 I conti 2007 si potrebbero chiudere con un minor gettito di entrate extratributarie di 3,6 miliardi, con una conseguente riduzione del "tesoretto" stimato nella Nota di aggiornamento da 5,9 a 2,3 miliardi. E non è finita qui! il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nel corso di un'altra audizione in Senato ha posto l'accento su come il contenimento della spesa primaria sia il problema centrale della finanza pubblica italiana e su come non si sarebbe fatto abbastanza nella manovra 2008. Il giudizio è negativo sulla finanziaria perché non sfrutta il favorevole andamento delle entrate per accelerare la riduzione del debito: non restituisce cioè ai contribuenti una quota significativa degli aumenti di gettito. Per Draghi «i progressi nella riduzione degli squilibri di bilancio sono modesti» e con la destinazione del "tesoretto" non al ripiano del *deficit* si metterebbe a rischio l'obiettivo del pareggio di bilancio. Non c'è peraltro neanche un taglio consistente sulle tasse dei lavoratori e delle imprese. Non c'è un freno alla dinamica della spesa pubblica, negli ultimi anni cresciuta ad un tasso reale del 2-2,5 Pertanto, la manovra 2008 comporterà secondo Bankitalia «un aumento netto delle spese di quasi 4 miliardi rispetto al tendenziale» e queste dinamiche «sono difficilmente compatibili con gli obiettivi di medio termine delineati nell'aggiornamento del DPEF». Tra le tante cose non previste da questa finanziaria, c'è la mancata eliminazione del *fiscal drag*. Così che anche gli sconti sull'ICI e sugli affitti previsti in finanziaria, di cui il Governo è andato tanto fiero, rischiano di essere negativamente compensati dal drenaggio fiscale. Vorrei intervenire sulla mia terra, sulla Calabria e sul Mezzogiorno. In questa parte del Paese il Governo ha preso tanti voti, la grande messe di voti non è stata utilizzata per risollevare le condizioni economiche

imbelle, sordo a tutte le aspettative delle popolazioni amministrate.

soltanto a focalizzarne due, forse marginali, inerenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, strategica a vario titolo. Il primo la soppressione dei contingenti di benzina agevolata, sinora goduti nelle Province di Trieste e Gorizia e da 25 Comuni della Provincia di Udine. Nessuna attività del Governo al riguardo per difendere tale regime è stata attuata in sede europea e del pari nessuna attenzione è stata dedicata per soluzioni compensative in una situazione economica di questa Regione particolarmente delicata. la Repubblica di Slovenia sta entrando in Europa con una serie di ricadute, ovviamente non positive, per l'economia di questa Regione di confine. La seconda tematica inerisce l'antico tema degli esuli istriani, il Governo aveva istituito un tavolo presso la Presidenza del Consiglio con la prima riunione tenutasi addirittura il 20 febbraio tra il Governo e le associazioni degli esuli, dove si era promessa una attenzione particolare per risolvere finalmente, con una nuova legge, il problema degli indennizzi e correlate tabelle fornite ed esaminate da codesto tavolo. Non vi è traccia di questa nuova legge nella finanziaria. Del pari una richiesta piccolissima che era stata garantita, cioè una interpretazione autentica per la rivalutazione degli assegni spettanti ai profughi, tema da affrontare con l'INPS, non solo non ha trovato soluzione positiva come era stato promesso, ma addirittura allo stato si è giunti ad una soluzione radicalmente opposta.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo e successivamente voteremo il disegno di legge finanziaria 2008, un provvedimento che rappresenta l'ennesima dimostrazione di come questo Governo gestisca maldestramente le risorse pubbliche e soprattutto senza nessuna precisa finalità economica e prospettiva di sviluppo. Il Governo ha infatti strutturato questa manovra economica preoccupandosi ancora una volta soltanto di tenere unita la sua maggioranza politica, piuttosto che indirizzarsi verso i reali interessi del Paese. Questa è una finanziaria *bluff*, l'ennesimo inganno per l'Italia e per gli italiani. In un sol colpo riuscite nell'intento di aumentare contemporaneamente spese e pressione fiscale, facendovi scudo, da un lato, con iniziative demagogiche e, dall'altro, distribuendo mance a pochi prescelti solo per rastrellare quelle esigue briciole di consenso che ancora vi sono rimaste. Colleghi, non è pensabile una visione così elastica dei conti pubblici, allentati o tirati da una parte e dall'altra, a seconda di chi fa la voce più grossa o di chi garantisce o meno il voto al provvedimento. Non è pensabile realizzare consistenti risparmi in quei settori che in tutti i Paesi avanzati vengono considerati strategici, come la ricerca, l'università, le infrastrutture, la sicurezza, la sanità, e stanziare invece ingenti risorse per ammorbidire le posizioni di qualche senatore. Come è possibile che mentre tra le famiglie italiane crescono numericamente i nuovi poveri voi vi occupate di foraggiare i fedeli amici e di programmare piccoli interventi *spot*? E quando il ministro Padoa-Schioppa afferma che le opposizioni fanno dell'allarmismo ingiustificato, viene da pensare che probabilmente vive in un altro Paese o evita di prendere in considerazione la difficile situazione delle famiglie italiane, che si sono viste recapitare una vagonata di aumenti sui generi di prima necessità, sull'acqua, sul gas, sull'elettricità; gente in condizioni disperate; salari inadeguati, pensioni da fame e nessuna risposta da questo Governo e da questa finanziaria. Il processo di riequilibrio avviato dal presidente Berlusconi è stato totalmente azzerato per far posto alle vostre logiche clientelari. D'altronde, colleghi, riuscire in così poco tempo a scontentare e deludere tutto e tutti è davvero un record. In tutti i settori, fra i dipendenti pubblici e quelli privati, tra i professionisti e i lavoratori atipici, fra gli operai e gli autonomi, cresce l'insofferenza l'insofferenza per le politiche vessatorie che stanno caratterizzando questi due anni di Governo. A ciò va aggiunto il coro unanime di critiche che arrivano dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali, dall'Unione Europea, alla Banca mondiale, al Fondo monetario internazionale, passando per le principali agenzie di *rating* finanziario, è all'unisono lo stuolo di giudizi negativi sull'operato di questo Governo. Così come sul fronte interno non vanno dimenticate le criticità più volte espresse dalla Corte dei conti e dal governatore della Banca d'Italia Draghi, che hanno denunciato la pericolosità per il Paese della politica economica del professor Prodi e compagni. Abbiamo una finanziaria mielosa, un Governo impantanato, perennemente rissoso nelle sue componenti, che cede ora ai ricatti delle sinistra radicale, ora alle pressioni delle piccole componenti non meglio collocate ed è più orientato a perseguire politiche di bandiera rispetto agli interessi visibili del nostro Paese. Davanti allo stato di disagio e di insicurezza che avvertono i cittadini italiani a causa della delinquenza dilagante e dell'allargamento delle maglie dell'immigrazione, voi sbandierate il tanto chiacchierato pacchetto sicurezza, salvo poi dimenticarvi che la gente non si sente più sicura neanche a casa propria e che le nostre Forze dell'ordine non hanno neanche i soldi per la benzina delle auto di servizio. Davanti al grido di dolore delle campagne italiane, all'importante e strategico ruolo svolto dai nostri agricoltori e allevatori, voi usate la mannaia e lasciate morire le nostre aziende sotto una montagna di debiti, mettendo in campo politiche deboli ed inefficaci. Così come, da sardo, mi preme evidenziare il fatto che nel luglio del 2009 l'isola di La Maddalena ospiterà un evento di importanza mondiale come il G-8 e che, a poco più di due anni, non si vede traccia di interventi destinati a trasformare il *summit* in una grande occasione di crescita per il territorio, infrastrutturandolo e mandando in vetrina uno dei poli ambientali più belli del Mediterraneo. Così come non vengono neanche previste le adeguate coperture finanziarie volte a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento sia per la popolazione locale che per quella ospite. Colleghi, gli italiani hanno provato sulla loro pelle gli effetti delle politiche economiche di Palazzo Chigi e di Padoa-Schioppa, una politica che toglie all'Italia l'ossigeno indispensabile allo sviluppo. Sono certo che anche in occasione di questo disegno di legge molti colleghi della maggioranza si troveranno in imbarazzo nel momento del voto e che, forse, solo lo spirito di lealtà verso il Governo o meglio la paura di perdere lo scettro del potere e il loro *status* li convincerà a votarla. Così come sicuramente troverà l'appoggio di alcuni di quei senatori che qui siedono per diritto di rappresentanza, per i grandi meriti raggiunti e che oggi sono costretti a «mercanteggiare» pochi spiccioli a sostegno di qualche loro iniziativa in cambio del loro voto. Assistiamo tra l'altro alla mortificazione del ruolo di qualche senatrice che oltre a svolgere i compiti istituzionali che le competono sono costrette a trasformarsi in «badanti» per paura di non mandare sotto il Governo. Preannunciando il mio voto contrario e quello del gruppo di Forza Italia al provvedimento in discussione, rivolgo un appello, e concludo Presidente, a quei senatori moderati che vivono costantemente in uno stato di disagio e che hanno recepito il malessere diffuso nell'opinione pubblica. Prendetevi la responsabilità di staccare la spina ad un Governo agonizzante. Un Governo che non modernizza il Paese, anzi lo arretra. Un Governo che non integra il Paese con l'Europa, anzi lo isola. Un Governo che non promuove la nostra economia, anzi soffoca le nostre imprese. Un Governo che assume per chiamata diretta, anziché per concorso. Un Governo che oggi dice di voler ridurre i componenti di Governo, dopo essersi prima opposto e poi averli moltiplicati. Speriamo, nell'interesse del nostro che si possa voltare pagina. Il primo è relativo all'economia reale ed alla crescita della ricchezza nazionale. La produttività del lavoro e dei fattori è tornata a crescere dopo anni di stagnazione o di arretramento, ma ad un ritmo che non appare in grado di farci recuperare l'enorme terreno perduto. In questo contesto, l'evoluzione del livello dei consumi interni ci propone, in tutta la sua cruciale portata, la cosiddetta questione salariale. Le politiche pubbliche (questo mi pare il problema), la politica economica possono qualcosa per affrontare e risolvere la questione salariale? Se possono qualcosa, questa legge finanziaria, così come esce dalla lettura della Commissione bilancio del Senato, muove nella giusta direzione oppure la contraddice? Il secondo Il secondo problema che voglio affrontare è relativo alla finanza pubblica e agli effetti delle modifiche della legge finanziaria approvate in Commissione; non sarebbe stato meglio, si è e ci ha chiesto il senatore Vegas ieri sera, utilizzare i risparmi di spesa definiti in Commissione (intanto registriamo che il senatore Vegas, a differenza di altri, registra che i risparmi di spesa in Commissione sono stati definiti e non sono pertanto inventati) non per finanziare nuova spesa, ma per ridurre il prelievo su famiglie ed imprese? Cercherò di dimostrare che è esattamente quello che abbiamo fatto. Sulla questione salariale, i punti di riferimento sono presto definiti. il primo, abbiamo salari e stipendi mediamente più bassi di quelli francesi del 20-25 per cento. Volutamente non scelgo la Germania, Paese ad altissima produttività del lavoro, dove la questione si pone in termini diversi, ma scelgo la Francia in quanto il paragone è più corretto. punto, alla base di questo andamento dei salari e degli stipendi c'è la mancata crescita della produttività. L'occupazione aumenta ed aumenta in modo significativo ormai da anni, in concomitanza con una debole crescita del prodotto. Questo significa che, siccome la produttività è il prodotto diviso il numero degli addetti, la produttività naturalmente si abbassa. Per affrontare il problema bisogna, dunque, agire contestualmente su tre terreni. Ripeto, agire contestualmente su tre terreni. bisogna favorire una contrattazione tra le parti protagoniste del conflitto sociale tale da redistribuire, anche a favore dei lavoratori, i vantaggi degli aumenti di produttività. La ristrutturazione dell'apparato produttivo del Paese nelle medie e grandi aziende è avvenuta. Ci sono vantaggi di produttività. Bisogna che avvenga una redistribuzione di questi vantaggi anche a favore dei lavoratori. Oggi non avviene. occorre rimodulare la pressione fiscale sui salari e gli stipendi in modo da innalzare il reddito disponibile delle famiglie e, in particolare, da premiare gli sforzi di incremento della produttività. bisogna investire sul capitale umano così da innalzare le potenzialità di crescita del sistema nel lungo periodo. Colleghi, in Commissione bilancio - non ne parla nessuno perché, secondo me, delle cose serie in realtà non si riesce mai a parlare a parlare - si è approvato un emendamento al comma 4 dell'articolo 1 che fissa per il Governo, nel 2008, un obiettivo molto chiaro: detto anno ci sarà un incremento del gettito superiore alle attese e alle previsioni incorporate nel bilancio a legislazione vigente, quel *surplus* dovrà essere usato per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. Dice così l'emendamento approvato.

Per i lavoratori autonomi in maggiore difficoltà, quelli delle imprese cosiddette marginali, la legge finanziaria dispone subito, e non in attesa della verifica dell'extragettito, interventi di straordinaria efficacia, a partire da quello che va sotto il nome giornalistico di forfettone. No, la scelta del comma 4 va letta in rapporto non ad un pregiudizio ideologico, bensì all'analisi che ho appena svolto sulla questione salariale: la produttività e l'esigenza di favorire una contrattazione che redistribuisca, a favore dei lavoratori dipendenti, i vantaggi di produttività che finalmente si stanno nuovamente determinando. E questa scelta è strettamente correlata a quella contenuta non nella finanziaria ma nel collegato *welfare*, relativa alla riduzione della pressione fiscale sulle quote di salario da premi di produttività. Intendiamoci: è l'avvio di un percorso e non il conseguimento della meta.

il patto del 1993, che ha svolto una funzione essenziale per il risanamento e il rilancio del Paese, ma che ormai ha perso quella che - con un gergo antico - si potrebbe chiamare la sua spinta propulsiva. In questo contesto leggo la scelta operata dalla maggioranza in Commissione bilancio in tema di *ticket* sulla diagnostica, di ICI sulla prima casa, di detrazione per il mutuo prima casa, di tassazione del gasolio da riscaldamento e di GPL nelle zone di montagna, di credito d'imposta automatico per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno; un credito d'imposta, signor Presidente, che sarà molto più alto nel 2008 (se il testo approvato in Commissione bilancio verrà definitivamente approvato ed entrerà a far parte della legge finanziaria) nel Mezzogiorno per l'assunzione di una donna rispetto all'assunzione di un uomo. Non è un cedimento al politicamente corretto, come qualcuno ha scritto. No, è il frutto della consapevolezza che noi abbiamo che innalzare la partecipazione delle donne alle forze di lavoro è uno dei due fondamentali pilastri di una politica di rilancio dello sviluppo. Se non alzeremo la partecipazione delle donne alle forze di lavoro, non otterremo questo risultato e, in funzione di questo, abbiamo fatto una norma che non ha precedenti nella storia - credo - della politica economica di alcun Paese europeo. Abbiamo differenziato un incentivo esplicitamente in nome dell'assunzione di donne al posto di uomini. Quello che ho appena fatto, colleghi, è l'elenco delle misure di maggiore impatto finanziario introdotte dalla Commissione bilancio nella legge finanziaria, così come consegnata dal Governo. Non sfugge a nessuno che sono misure che, comprensivamente, valgono molto più di un miliardo e mezzo di euro

non abbiamo approvato nemmeno una norma di aumento delle aliquote delle basi imponibili rispetto al testo del Governo. Le coperture sono tutte assicurate o da riduzioni di spesa o da utilizzo di risorse tabellari senza praticare nessun'altra copertura. Si poteva fare di più sul lato della riduzione della spesa? Se il principale e più autorevole quotidiano economico del Paese continua a confrontare il risparmio scritto dalla Commissione bilancio nella legge finanziaria con le dichiarazioni di un Ministro, quali ovviamente non vi è traccia nella relazione tecnica della legge finanziaria stessa, io dubito che si possa cercare di rispondere seriamente a questa domanda.

Non sono affatto persuaso, infatti, degli argomenti portati dal Ministero dell'economia per ridurre i risparmi attesi dal rilancio della CONSIP nella sua funzione originaria (così come alla fine come alla fine degli anni Novanta), né dagli argomenti addotti dallo stesso Ministero per ridimensionare i tagli delle spese per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili pubblici o per ridimensionare gli aumenti attesi di entrate ottenibili da quella stessa fonte. modo, resto convinto del fatto che un ben organizzato piano per accorpare e razionalizzare in tre anni tutti gli uffici periferici dello Stato centrale possa, al tempo stesso, migliorarne le *performance* e ridurre la spesa. Nei prossimi mesi, riaffronteremo l'argomento. Una cosa, però, è già certa: dal versante della riduzione dei costi impropri della politica, quei significativi risparmi - non compresi nel disegno di legge originario del Governo arrivato al Senato, così come dimostra la relazione tecnica

*(RC-SE)*. Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, la mia parte politica considera questa finanziaria 2008 un un importante passo avanti verso politiche innovative su questioni relative a politiche sociali, alla lotta al precariato, alle affermazioni del diritto al lavoro, alle politiche ambientali.

dal Governo in termini politici, ma che questo stenta a riaffermare in sede di finanziaria e di allocazione di risorse finanziarie. Vorrei parlare anzitutto di cooperazione internazionale, del tema della riduzione delle spese militari e della riconversione dell'industria bellica. sottolineare, con molta soddisfazione, che il decreto sull'extragettito ha permesso al Governo di colmare alcune gravi e importanti lacune e ritardi nell'assolvimento di impegni internazionali relativi alla cooperazione internazionale, alla partecipazione italiana alle Agenzie multilaterali delle Nazioni Unite e alla lotta alle grandi pandemie. Su questo ultimo punto vorrei ricordare che almeno 130 milioni di euro sono stati stanziati per pagare la rata del 2008, dopo aver già provveduto a stanziare le cifre necessarie al risanamento degli arretrati sulle altre rate mai pagate, per un totale di 260 milioni di euro. Altro importante contributo viene stanziato per le banche multilaterali di sviluppo, tra cui la Banca mondiale. E proprio in quella sede la Commissione affari esteri del Senato ha avuto occasione di riaffermare alcuni impegni già assunti dal Governo con degli ordini del giorno approvati in quella sede, che tra l'altro impegnano il Governo ad opporsi, o comunque a sostenere una moratoria a sostegno di politiche di privatizzazione dei beni comuni e dell'acqua da parte di queste banche multilaterali, e anche a procedere alla revisione delle condizionalità di accesso a programmi di riduzione e cancellazione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo. Il tema del debito estero è toccato in finanziaria nell'articolo 48, con il capitolo relativo, appunto, al supporto a programmi di cancellazione del debito multilaterale, ovverosia del debito dei Paesi in via di sviluppo verso le istituzioni finanziarie e multilaterali (in terminologia tecnica MDRI) e al supporto degli obiettivi di sviluppo del millennio, a programmi per nuovi meccanismi innovativi per il finanziamento dello sviluppo. Proprio su questo va riconosciuto che il Governo, in particolare il Ministero degli affari esteri, ha già assunto una serie di impegni molto importanti, decidendo di partecipare a differenza del passato - al gruppo di Rio, che sta lavorando a programmi di finanziamento innovativi in vista del vertice di Doha del 2008, nel quale si farà il punto sull'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza ONU di Monterrey del 2002 sulla finanza per lo sviluppo. In questa occasione vorremmo chiedere al Governo di impegnarsi a partecipare anche al gruppo di lavoro *ad hoc*, previsto appunto per il processo che porterà a Doha e che dovrebbe studiare meccanismi di tassazione innovativa a livello globale per finanziare, appunto, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. La Commissione affari esteri del Senato ha poi approvato un ordine del giorno, accolto e sostenuto anche dal Governo, che prevede la creazione in tempi rapidi di una Commissione di studio e di analisi sul debito estero dei Paesi in via di sviluppo, o meglio sulla situazione creditizia dell'Italia verso quei Paesi, al fine di determinare la qualità, l'efficacia, l'efficienza (mi permetto di aggiungere anche la legittimità) dei crediti concessi, dei debiti contratti da quei Paesi, considerandone gli aspetti legali e finanziari, nonché quelli economici, sociali ed ambientali. L'emendamento che abbiamo presentato è stato dichiarato inammissibile, però io credo che quell'ordine del giorno, approvato con il sostegno di tutte le parti politiche in Commissione, costituisca un impegno verso il Governo affinché questa Commissione venga istituita per contribuire al dibattito internazionale sul debito e sulla trasparenza del debito estero, ed anche per rafforzare i princìpi della corresponsabilità dei creditori verso quei Paesi e i mercati finanziari internazionali.

quindi, che sia un impegno coerente rispetto a qualcosa che era già stato fatto in passato, soprattutto per quanto riguarda lo studio sui processi di riproduzione del debito estero e su come il debito estero e i meccanismi di cancellazione o riduzione dello stesso oggi possano impattare positivamente o negativamente nel perseguimento di obiettivi di sviluppo del millennio. Vorrei ricordare che tra questi obiettivi di sviluppo ce n'è uno che riguarda la cooperazione internazionale e che impegna i Paesi firmatari, tra cui anche l'Italia, a raggiungere entro il 2015 la quota dello 0,7 per cento del PIL da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo. Su questo va sottolineato, purtroppo, un grave ritardo. Nonostante l'ultimo DPEF prevedesse un tragitto che dovrebbe accompagnare il nostro Paese verso il perseguimento dello 0,55 per cento del PIL come obiettivo intermedio entro il 2008, la finanziaria, con gli con gli stanziamenti in tabella C, non sembra recepire questi indirizzi, né, appunto, sembra tener conto appieno degli impegni che l'Italia ha assunto verso la comunità internazionale: impegni che riguardano non soltanto l'aspetto quantitativo, ma anche quello qualitativo. Tra l'altro, la Commissione affari esteri del Senato è chiamata in questo periodo a discutere la riforma della cooperazione internazionale. Devo sottolineare che ci stiamo trovando in un momento di difficoltà nel procedere con questo processo di discussione nel Comitato ristretto e vorrei anche sottolineare con altrettanta con altrettanta evidenza come questa discussione è seguita molto attentamente all'esterno dalle organizzazioni non governative italiane, dalla società civile, dall'ONU e dell'OCSE, che proprio l'anno prossimo dovrà svolgere una valutazione della cooperazione italiana allo sviluppo. Insomma, alcune occasioni sono state mancate, ma noi ci ripromettiamo di continuare a lavorare insieme alla società civile italiana e internazionale, insieme al Governo ed anche in questa maggioranza, affinché queste occasioni vengano finalmente riprese e venga dato un seguito coerente alle politiche, appunto, del Governo. Vorrei ricordare i 30 milioni stanziati per il G8 del 2009 alla Maddalena. Già in Commissione affari esteri abbiamo avuto occasione di sottolineare come la formula del G8 sia oramai vetusta, obsoleta, non risponda più a quegli obiettivi di democratizzazione della *governance* globale che pure il nostro Governo vuole sostenere a livello di Nazioni Unite. In questa occasione chiediamo

che rientri nell'alveo delle Nazioni Unite e permetta veramente la costruzione di un sistema di *governance* globale democratico e multipolare. In conclusione del mio intervento mi soffermo sul tema delle spese militari e della riconversione dell'industria bellica.

Costituzione, che veda nella diplomazia, nella mediazione, nella prevenzione civile dei conflitti i suoi cardini essenziali e che stentiamo a credere possa essere assolta da sistemi d'arma sofisticati dalla marcata connotazione offensiva, come ad esempio lo *Joint straight fighter* o altri sistemi d'arma che verranno finanziati in questa legge finanziaria. Ridiscutere le spese militari e la riconversione dell'industria bellica significa per noi anzitutto ridiscutere gli strumenti militari della nostra politica estera, fare chiarezza sull'intreccio tra interessi dell'industria e strategie militari del nostro complesso industriale militare e sostenere politiche industriali di riconversione che non siano penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici ma che siano senz'altro coerenti con strategie politiche, produttive e industriali che mettano al centro l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la dimensione civile della sicurezza a livello nazionale e internazionale. È un processo certamente difficile, lungo, ma ineludibile per dare rappresentanza ad ampi settori della società civile e dell'opinione pubblica e anche sindacale italiana,

Essa si presenta con provvedimenti che vanno nella giusta direzione e coniugano equità sociale con sviluppo di qualità. È evidente che tale giudizio si riferisce al testo al nostro esame,

Il giudizio finale ci riserviamo di esprimerlo nella dichiarazione di voto finale. Si è sostenuto, in queste settimane, che la finanziaria è troppo "timida" nei tagli alla spesa pubblica. Si sta alla spesa pubblica. Si sta riproducendo la discussione avvenuta durate i lavori per l'approvazione del DPEF. In verità non si tiene conto che: 1) Il programma di rientro dal *deficit* ("*deficit* zero") è stato mantenuto e si completerà come da impegno con l'Unione Europea entro l'anno 2011. Rispetto a poco più di un anno fa le finanze pubbliche italiane sono pienamente tornate sotto controllo. Dopo quattro anni consecutivi di sforamento dei parametri europei, nel 2007 il disavanzo pubblico è finalmente rientrato sotto la soglia del 3 per

2) Nel 2007, a fronte di una pressione fiscale salita di 0,8 punti (a parità di aliquote e esclusivamente grazie al recupero di evasione), le spese correnti primarie sono rimaste immutate al 39,9 per le maggiori entrate si sono tradotte in un aumento dell'avanzo primario; nella scorsa legislatura la spesa corrente primaria è cresciuta inesorabilmente anno dopo anno dal 37,3 per cento del 2000 Ridurre progressivamente e soprattutto riqualificare le nostre spese pubbliche, rendendole più rispondenti alle esigenze di lavoratori, famiglie e imprese, costituisce un obiettivo centrale; l'intervento sui residui passivi (le somme non spese) previsto dalla finanziaria - che affronta una delle questioni centrali della capacità di spesa effettiva delle amministrazioni, sottolineata dalla presenza nel bilancio pubblico di residui passivi per decine di miliardi di euro - comporta una riduzione strutturale dei volumi di spesa. 3) L'attuale congiuntura vede una diminuzione delle previsioni di crescita e non aiuterebbe certo al Paese un taglio eccessivo della spesa pubblica. pubblica. 4) Si tagliano e si razionalizzano qui, diverse voci di spesa per un totale di 3.720 milioni nel 2008 per arrivare a più di 4 miliardi nel 2010.

Una manovra, per questa sessione di bilancio, complessa ed articolata, che si presenta con la Nota di aggiornamento al DPEF e con il bilancio diviso in 34 missioni. Sottolineo l'importanza di questo fattore che rende più trasparente e più leggibile il bilancio stesso,

ai singoli Dicasteri di spesa e parte dalle missioni e dai programmi per poi saldarsi ai centri di responsabilità. Un bilancio che stanzia risorse aggiuntive rispetto al 2007: 1800 milioni di euro in più per "competitività e sviluppo delle imprese", 160 milioni di euro in più per "soccorso civile", 265 milioni di euro in più per "istruzione scolastica", 420 milioni in più per "l'Italia in Europa e nel mondo", 3.100 milioni in più per "politiche previdenziali", 320 milioni in più per "diritti sociali, solidarietà, famiglia", 70 milioni in più per "immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", 6.700 milioni più per relazioni finanziarie con le autonomie territoriali". La finanziaria oggi al nostro esame, facendo leva sul minore *deficit* della finanza pubblica, presenta una manovra leggera di appena 11 miliardi, coerentemente con il DPEF approvato lo scorso luglio. Presenta, inoltre, un decreto-legge contenente misure urgenti di finanza pubblica, già discusso ed approvato da questa Assemblea, un collegato cosiddetto di "sessione" da approvare entro il 31 dicembre, che recepirà i contenuti del protocollo su *welfare e* lavoro sottoscritto il 23 luglio scorso e che è in prima lettura alla Camera dei deputati,

Avevamo chiesto unitariamente (assieme ai Gruppi Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) che il Consiglio dei ministri varasse una manovra finanziaria per il 2008 che assumesse le priorità che erano alla base del programma dell'Unione e del nostro impegno con gli elettori, primo fra tutti l'equità sociale. Innanzitutto la questione salariale, se è vero com'è vero - è stato ricordato appena qualche minuto fa dal presidente Morando - che i salari medi nel nostro Paese sono mediamente più bassi rispetto ad altri Paesi europei importanti come l'Italia (non siamo solo noi a dirlo, lo dicono tutti, compresi il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente di Confindustria) e se è vero come è vero - ormai è patrimonio di tutti - che negli ultimi, a fronte di una diminuzione del valore del lavoro e del potere di acquisto dei salari si è registrata, invece, una crescita delle rendite e dei profitti. Pertanto, si rendono necessarie una serie di politiche volte a riequilibrare i rapporti tra salari, rendite e profitti. Avevamo chiesto maggiore tutela dell'ambiente e adeguate misure per far fronte ai cambiamenti climatici, la lotta alla precarietà del lavoro, maggiori investimenti nei settori strategici per il futuro del Paese, un impegno ulteriore nella lotta all'evasione fiscale e contributiva, l'adeguamento della tassazione delle rendite, un intervento deciso in materia di riduzione dei costi della politica e una più incisiva lotta agli sprechi e all'uso delle risorse Un complesso di interventi, per i quali abbiamo formulato proposte di spesa ma anche l'individuazione delle risorse necessarie per attuarle, consci che occorre fare molto di più: per l'applicazione del Protocollo di Kyoto, per promuovere una politica energetica basata su fonti energetiche rinnovabili; per sostenere interventi di risparmio ed efficienza energetica nel campo dell'edilizia; per il potenziamento del trasporto pubblico sostenibile nelle città; per attuare una forte azione contro la precarietà a partire da ciò che l'ha generata strutturalmente, ovvero i contratti di formazione lavoro; per invertire la tendenza negativa che, in questi anni, ha portato ad una compressione della spesa sociale e che ha prodotto nuove insicurezze e povertà. Un primo passo in questa direzione era già stato segnato con il decreto-legge n. 81 del luglio scorso (ora legge n. 127 del 3 agosto 2007), nel quale si provvedeva a: aumentare le pensioni di importo basso,

bonus per gli incapienti, e famiglie più deboli per un milione e 900.000 euro; un piano casa per 550 milioni per assicurare la casa alle fasce più deboli della popolazione; interventi per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per 70 milioni; interventi in materia di energie rinnovabili; interventi per ricerca e formazione 500 milioni; interventi per infrastrutture e azione di sviluppo 2 miliardi; la moratoria dei processi di privatizzazione dell'acqua, a difesa dell'interesse primario per il genere umano, per sottrarlo ad ogni possibile speculazione o interesse di parte, perché l'azione pubblica difenda e valorizzi uno dei beni più preziosi, l'elemento che determina la vita del pianeta; il rilancio del ruolo di pace dell'Italia e delle attività di cooperazione internazionale con uno stanziamento di ulteriori 900 milioni, per citare solo alcuni dei principali titoli contenuti nel decreto-legge, che abbiamo recentemente approvato. La finanziaria La finanziaria 2008, continua lungo questo sentiero e già nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, presenta elementi sostanziali di novità, soprattutto in termini di trasparenza e snellezza, occorre sottolineare che rafforza il segno intrapreso l'anno scorso: il risanamento della finanza pubblica che ha acquisito qui carattere di strutturalità. Non si tolgono risorse, non si presentano tagli drastici, si prosegue nell'opera di riqualificazione della spesa pubblica introducendo elementi di redistribuzione del reddito. non vengono ridotti i capitoli riguardanti lo Stato sociale e non si interviene sulle spese degli enti locali (come purtroppo è avvenuto negli anni passati), limitandosi ad aggiustamenti nella conduzione delle regole del Patto di stabilità interno e premiando i Comuni e gli enti locali virtuosi. di legge finanziaria, nel testo approvato dalla Commissione bilancio dopo un lungo lavoro svolto unitariamente dalla maggioranza, presenta ulteriori significativi aspetti positivi e migliorativi, che spero vengano mantenuti fino alla fine. Per tali risultati sottolineo il forte impegno propositivo svolto dalle senatrici e dai senatori del nostro Gruppo e di tutti i Gruppi della Sinistra.

tale unità di progetti nasce e si verifica non su astratte formulazioni, ma sulle risposte da dare al Paese, a partire dai bisogni espressi dai lavoratori e dagli strati popolari. un progetto e di un lavoro avviato nelle istituzioni, non affidato soltanto alle iniziative dei gruppi dirigenti dei partiti che li rappresentano nelle istituzioni, ma che guarda ad una nuova prospettiva: la partecipazione diretta ed ampia dei militanti, degli elettori e dei cittadini, delle donne e degli uomini, che non si rassegnano a seppellire la storia e l'idea di una sinistra politica italiana. Tale progetto trova sostanza e verifica nel lavoro unitario che si sviluppa nei territori e nelle Regioni: un percorso unitario che avrà un importante primo approdo, per delineare il percorso comune, nell'iniziativa unitaria che si terrà a Roma l'8 e il 9 dicembre prossimi. Il grande lavoro svolto dalla Commissione bilancio - frutto anche dell'impegno e della competenza del presidente Morando e della capacità dei relatori Legnini ed Albonetti e dell'impegno profuso con serietà e potenza da tutti i componenti della Commissione, in particolare della maggioranza - ha evitato per il prossimo anno il ritorno dei *ticket* sanitari sulla diagnostica. Si tratta di un intervento che comporta oneri a carico del bilancio dello Stato per circa 850 milioni di euro. Trovo del tutto strumentale la polemica in ordine alla copertura. Dà una definitiva risposta al precariato nella pubblica amministrazione prevedendo la realizzazione di piani triennali che operano per il progressivo passaggio a tempo indeterminato di tutti coloro che da anni sono impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Anche qui non capisco le critiche rivolte a questa parte della legge oggi al nostro esame. Si tratta di interventi di giustizia e di equità utilizzati, in aggiunta, altre volte dal Parlamento anche per altri settori della pubblica amministrazione. Mi riferisco, per esempio, alla scuola.

superando in tal modo anche il dramma che esiste in molte aree del Mezzogiorno, dove troppi lavoratori perdono il lavoro quando sono ancora troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per poter essere reimpiegati specie a fronte di meccanismi che incentivano altri tipi di rapporto di lavoro. L'incentivo viene concesso a patto che le aziende siano in regola con le norme in materia di sicurezza, che non abbiano proceduto a licenziamenti nel periodo immediatamente precedente, che si impegnino a conservare i posti di lavoro creati per almeno tre anni. Si tratta di incentivi differenziati secondo il genere. Su questo non aggiungo nulla rispetto a quanto appena detto dal senatore Morando. Per far fronte al fenomeno del caro mutui si innalza del 10 per cento il tetto di detraibilità delle spese per interessi sui mutui prima casa, portandolo a 4.000 euro. La nostra proposta era di elevarlo a 5.000 euro, ma intanto quello ottenuto è un risultato. Ha eliminato il tetto di reddito per usufruire della detrazione ICI per la prima casa, mentre si escludono le abitazioni di lusso; si reintroduce la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza degli asili nido. Per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, ovvero composti solo da minori non inabili, vengono aumentati gli importi degli assegni familiari. Poi, anch'io penso che vada sottolineata come norma di particolare rilievo la previsione contenuta all'articolo 1, dove è previsto appunto che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e da una diversa politica economica del Paese che si realizzeranno nel 2008 vadano a ridurre la pressione fiscale sui lavoratori, aumentando l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente e per pensioni. Credo si tratti di una norma di straordinaria importanza. Viene introdotta tutta una serie di norme di salvaguardia dell'ambiente; in particolare, viene interamente riscritta la normativa in materia di energia da fonti rinnovabili e si prevedono incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti da adibire a trasporto pubblico locale. Si istituisce un fondo in favore di tutte le vittime dell'amianto o dei loro eredi che hanno contratto patologie correlate. Il fondo eroga un contributo economico aggiuntivo alla rendita diretta a favore dei superstiti che è già prevista dalla norma in vigore. Ancora, per i lavoratori autonomi e le piccole imprese (circa 900.000 contribuenti) si è operata una semplificazione degli adempimenti. Questo porterà una sensibile riduzione dei costi; inoltre, i contribuenti con un volume di affari sotto i 30.000 euro l'anno e che non hanno investimenti superiori a 15.000 euro negli ultimi tre anni avranno un'unica imposta da pagare pari al 20 per cento, che assolve a tutti gli obblighi (IVA, IRAP e IRPEF). Si consegue un grande risparmio in ordine ai costi burocratici. Si tratta, comunque, di una misura che il contribuente, se rientrerà nei parametri e vorrà, potrà scegliere per adempiere ai suoi obblighi tributari, fermo restando il vecchio sistema se non dovesse, per diverse ragioni, convenirgli. È una norma che tiene conto di quanto sostenuto dai rappresentanti delle categorie del lavoro autonomo e che fa seguito alla sostanziale rivisitazione, già avvenuta in precedenza, delle altre norme a favore di queste categorie, in modo particolare degli studi di settore. Importanti e qualificati sono gli interventi in materia di energia, che consentono di procedere rapidamente alla diffusione delle energie alternative - come l'eolico, il fotovoltaico e le biomasse agricole nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Numerosi sono anche gli interventi introdotti in tema di salvaguardia ambientale: dalla realizzazione di aree verdi urbane, alla prevenzione del rischio idrogeologico, agli incentivi per sviluppare nuove tecnologie del del riciclaggio e smaltimento del rifiuto, al potenziamento delle aree marine protette. Sono stati introdotti strumenti innovativi di controllo e di intervento per fronteggiare anomali incrementi dei prezzi dei prodotti alimentari; si è dato impulso allo sviluppo e alla diffusione dei cosiddetti GAS (Gruppi di acquisto solidale), chiarendo il regime fiscale di attività di acquisto collettivo. Resta aperta la grande questione della tassazione delle rendite finanziarie o, meglio, l'omogeneizzazione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie. Il Governo si è dichiarato d'accordo con la proposta della sinistra, ma ha addotto il motivo della complessità del problema per chiedere più tempo per presentare una proposta organica. Si è operato, tra l'altro, per ridurre significativamente il numero dei componenti del Governo, con il ritorno alla cosiddetta legge Bassanini, introdurre un tetto al trattamento economico per chiunque riceva, dalle pubbliche finanze, emolumenti o retribuzioni (su questo sarà più preciso il senatore Villone), per razionalizzare e qualificare le strutture, le aziende ed i consorzi, istituiti tra gli enti territoriali per la gestione di importanti servizi civili e sociali tra cui il ciclo integrato

a mia disposizione, mi avvio alla conclusione. Va tenuto presente che forse è la prima volta, grazie anche ai miglioramenti introdotti in sede di discussione in Commissione bilancio, che la manovra finanziaria, piuttosto che un coacervo spesso confuso di misure, assume la connotazione di una tappa nella realizzazione di un programma, dalla quale emerge il disegno, dai contorni ancora non ben netti e definiti, di un'Italia più giusta e più efficiente. Mi permetto di sottolineare che naturalmente è stato fondamentale il lavoro e l'atteggiamento unitario della sinistra, sempre teso a rafforzare il Governo e mai ad indebolirlo. Tutto ciò, come già sottolineato in apertura di intervento, motiva l'espressione di un giudizio positivo, da cui è dipesa la scelta del mio Gruppo di non presentare emendamenti per la discussione in Aula. Speriamo che tale giudizio possa essere mantenuto - ripeto - fino alla fine e che il testo al nostro esame possa essere approvato senza stravolgimenti o modifiche tali da alterarne l'indirizzo e la filosofia complessiva.

Il ministro Padoa-Schioppa ebbe a definire questa manovra come un progetto di ampio respiro, di ampie vedute, capace di guardare al futuro del Paese.

limitata e dimostra tutte le debolezze e i limiti di una coalizione di Governo incapace di creare prospettive serie per il nostro Paese. L'Italia ha bisogno di altro, non ha bisogno di improvvisazioni. L'Italia non ha bisogno di progetti determinati dai ricatti e dai condizionamenti di alcune forze politiche minori all'interno di questa maggioranza. L'Italia ha bisogno di affrontare i problemi strutturali interni al Paese

Ci sarebbe stato quindi bisogno di una politica importante, virtuosa, capace di imprimere un taglio di sicura incisività alla programmazione politica ed economica. Tutto ciò in realtà non è avvenuto,

che si ritroveranno sulle spalle le conseguenze delle mancate scelte di questo particolare momento storico. Noi comprendiamo perfettamente - lo diciamo in maniera molto franca agli esponenti del Governo esponenti del Governo - che nel momento in cui si adotta e si approva una legge finanziaria si creano le condizioni e i presupposti per subire i condizionamenti di alcune corporazioni, *lob**bies*, gruppi economici ben organizzati,

non toglie che quando un Governo ha idee ben precise sui propri paradigmi di sviluppo, crea le condizioni per resistere a questi condizionamenti che molte volte non producono assolutamente nulla di positivo ma, al contrario, le opportunità peggiori

Pertanto, di fonte ad una situazione di questo genere, credo che sia assolutamente necessario andare ad esaminare molto rapidamente, nello spazio di pochissime battute, tutte le vostre inadempienze e anche tutte le azioni che avete posto in essere per far apparire al Paese

forza ed intensità. Avete cercato poi di raggirare anche il sistema imprenditoriale quando avete sostanzialmente determinato le premesse per la diminuzione dell'IRES dal 33 per cento al 27,5 per cento da un lato, mentre dall'altro cambiava sostanzialmente tutta l'impostazione fiscale sugli accantonamenti e sugli interessi passivi per cui in una sorta di gioco delle tre carte toglievate con la mano sinistra quanto davate con mano destra. È un fatto assolutamente grave

una delle palle al piede più pericolose all'interno dell'intero sistema-Paese e pur tuttavia, senza aver modificato assolutamente nulla per accelerare i processi, ad iniziare da quelli tributari, avete creato le condizioni per proporre invece in finanziaria una misura volta a sopprimere l'arbitrato,

Mi auguro che sotto questo profilo vi sia un'ampia riflessione da parte di questo Governo, altrimenti le questioni da affrontare nei prossimi mesi saranno di una gravità inaudita e non sarà assolutamente possibile porvi rimedio.

Gli esempi sono due. Personalmente ho presentato un emendamento che allungava i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione; cosa che non è un frutto del Governo di centro-destra, ma è una delle pochissime iniziative positive che avevate adottato, sia pure in maniera raffazzonata, con il vostro Governo. Avete ritenuto di dire di no, di fatto non smentendo chi presentava e vi sottoponeva l'emendamento; piuttosto, la vostra azione di Governo, dimostrando in questa maniera che probabilmente è stato anche un fallimento quel tipo d'iniziativa che avevate assunto, così come avete lasciato un *vulnus* importante per quanto riguarda gli ispettori del lavoro. Non credo che si possano determinare le condizioni per sistemare l'intero sistema produttivo se non si creano i presupposti anche per un controllo efficace sul sistema produttivo medesimo. Ma la vostra inconsistenza è stata tale da porre in una situazione di secondo piano queste situazioni, così come è avvenuto per il sistema della sicurezza. Fuori di qui è in

infine, la penalizzazione del Mezzogiorno d'Italia, che non trova più sede nel dibattito politico del centro-sinistra, soprattutto dicendo chiaramente che che volete sfuggire al confronto parlamentare attraverso il voto di fiducia. Per quanto ci riguarda, avendo compreso perfettamente i vostri intendimenti, non vi permetteremo questo ulteriore insulto all'intelligenza del popolo italiano.

contiene ed affronta numerosi articoli riguardanti i trasporti, le infrastrutture e le regole di Governo di questo settore. È un segno concreto e positivo di una attenzione determinata ad un sistema oggi fortemente inefficiente ed inquinante, con la proposta di alcune misure positive, di cui parlerò, ma che registra su alcuni punti purtroppo ancora una evidente continuità con alcune scelte sbagliate del passato, senza indicare quelle necessarie soluzioni innovative per il futuro, in particolare per le infrastrutture che servono il nostro Paese. Partiamo dal tema delle città e della mobilità nei nostri centri urbani. Con questa manovra finanziaria, e positivamente, sono assegnati circa 500 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, per migliorare il servizio, la qualità dei mezzi e l'efficienza delle reti. Si tratta di risorse utili e certamente positive. Per la prima volta va anche sottolineato che la legge finanziaria contiene la defiscalizzazione degli abbonamenti nel trasporto locale, regionale ed interregionale, come forma di sostegno attiva a chi utilizza i mezzi collettivi: un ottimo risultato - lo voglio sottolineare - che risponde ad una richiesta decennale delle amministrazioni locali, delle imprese di trasporto e degli ambientalisti. Voglio al contempo sottolineare due criticità che persistono rispetto al Fondo per il trasporto pubblico locale: le risorse assegnate sono ancora insufficienti per superare la carenza cronica di offerta di servizi di qualità ai cittadini e, soprattutto, si tratta di un fondo previsto solo per l'anno 2008, quindi senza quel carattere stabile e duraturo che la situazione di inquinamento e congestione delle nostre città, invece, richiederebbe. Del resto, era stato lo stesso tavolo interistituzionale, istituito dal Governo presso la Presidenza del Consiglio con Federmobilità, (cioè le Regioni), ASSTRA (le imprese di trasporto) e le organizzazioni sindacali, ad indicare come soluzione strutturale un Fondo alimentato annualmente mediante il prelievo di una quota dell'accisa sul gasolio non professionale. Ma questa soluzione strutturale non è contenuta nella legge finanziaria 2008 e, proprio per questa ragione, il settore ha indetto per il 14 novembre 2008 una giornata di mobilitazione. A questa criticità va aggiunto il fatto che con questa manovra non vengono aumentate le risorse per il Fondo mobilità sostenibile, né per il Fondo pendolari, per l'acquisto di bus, tram e treni, entrambi istituiti con la legge finanziaria 2007. Abbiamo raccolto queste obiezioni che vengono alla manovra dal mondo delle città e delle imprese di trasporto e nella Commissione bilancio ci siamo fatti carico di presentare un apposito emendamento, cui il Governo ha però obiettato di non avere ancora una soluzione strutturale da inserire nella manovra, riconoscendo però che questo tavolo è aperto e che tale soluzione andrà individuata.

quella già prevista dalla finanziaria 2007 per l'annualità 2008) e 4,2 miliardi di nuove risorse per la legge obiettivo Ma i problemi, per il nostro Gruppo restano sia nella qualità della spesa per gli investimenti, sia nel mancato superamento della legge obiettivo. Infatti, ad oggi, il Governo non ha ancora presentato il promesso disegno di legge di riforma, come scritto nel programma dell'Unione e come sollecitato più volte dal Parlamento, anche, per esempio, in sede di espressione del parere sul DPEF nel luglio 2007. Ci aspettiamo, e lo vogliamo sottolineare anche in questa occasione, che, come indicato nella Nota di variazioni, il Governo, entro il 15 novembre, presenti un provvedimento su trasporti, infrastrutture ed assetti del territorio che contenga anche quei due o tre punti critici che il superamento della legge obiettivo richiede come soluzione, in particolare il ripristino della Conferenza dei servizi, sede in cui le istituzioni locali possono decidere le infrastrutture che interessano il loro territorio. Quindi, secondo il nostro Gruppo, le risorse sono ancora in misura troppo rilevante destinate alle autostrade, mentre gli investimenti sulle reti urbane, metropolitane e tranviarie non sono ancora presi in adeguata considerazione a causa del *deficit* che attanaglia le nostre città. Questi sono pertanto i punti maggiormente critici: il mancato superamento della legge obiettivo e le scarse risorse destinate alle città. Vorrei fare poi una specifica sottolineatura sul tema del federalismo infrastrutturale che anche con questa manovra, estendibile a tutte le Regioni italiane, viene proposto dal Governo in materia di strade, autostrade ed ANAS. I Verdi non sono affatto contrari all'idea di federalismo infrastrutturale, ma, con un apposito emendamento, purtroppo ancora non accolto, hanno prospettato un sistema di regole trasparenti e omogenee tra le diverse Regioni per gestire queste società all'interno di una strategia condivisa di politica dei trasporti e di scelta motivata della lista delle opere utili. Se da un lato è giusto avvicinare la decisione ai livelli più bassi ed ai livelli territoriali, coinvolgendo quindi anche le istituzioni locali (in questo senso è ancor più inaccettabile il mantenimento della legge obiettivo), tale quadro di regole in ordine ai concessionari ed alla scelta delle opere deve però essere realizzato in un ambito di massima trasparenza, cosa che purtroppo la norma non chiarisce e non fa. Infine, voglio ricordare che sempre in materia di investimenti la manovra prevede misure significative per la sicurezza stradale con circa 204 milioni di euro per il periodo 2008-2013; risorse decisamente maggiori rispetto alla finanziaria precedente, ma - lo voglio sottolineare - ancora non adeguate ad attuare il Piano per la sicurezza stradale del 1999. Per quanto riguarda i porti ed il settore marittimo, la manovra conferma la volontà del Governo di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, anche attraverso una quota, che le Regioni potranno trattenere, dell'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise derivate dalle operazioni nei porti. Misure di sostegno sono previste anche per l'industria cantieristica e le imprese armatoriali, nonché un incremento per il Fondo per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di aumentare complessivamente la sicurezza della navigazione, anche in correlazione agli incrementi dei dati di traffico.

destina complessivamente circa 366 milioni di euro; si tratta di obiettivi importanti di riequilibrio modale, ampiamente coerenti con l'impegno del Governo italiano a rispettare la battaglia contro l'effetto serra. Va anche sottolineato tuttavia che all'autotrasporto delle merci continuano ad essere destinate, anche quest'anno dalla legge finanziaria 2008, ingenti risorse pari a 313 milioni di euro che, se sommati a quelli previsti dalla

del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, un'evidente sproporzione tra le risorse destinate all'innovazione e al riequilibrio modale e quelle destinate all'autotrasporto. In conclusione, con questa manovra il Governo Prodi conferma il proprio impegno per i trasporti e le infrastrutture,

al ricordo di Enzo Biagi, scomparso questa mattina. Abbiamo avuto anche opinioni diverse con il collega in giornalismo Biagi, ma non c'è bisogno che io insista su quanto egli fosse bravo. Voglio soltanto lasciare una notazione a suo ricordo; quando scompare un giornalista, soprattutto quando è bravo, è come quando muore un giornale: viene meno una voce della libertà. È proprio in omaggio alla libertà che dedico questi pochi secondi al mio caro collega Biagi. Sarò brevissimo, per l'ora, ma anche perché il tempo che mi è concesso è poco; sette minuti non sono molti per affrontare un tema come quello della finanziaria e andrò quindi all'essenziale,

e poi un tema che da anni vado rilevando nei miei interventi parlamentari, di tornare cioè alla semplice legge di bilancio, mandando finalmente in soffitta la finanziaria, che è una legge che ha complicato molto i problemi del bilancio dello Stato e fatto sì che essi si configurassero come una sorta di mercato delle vacche; un'espressione usata

«Nel complesso, la manovra accresce l'indebitamento netto del 2008 di 6,5 miliardi. Essa reperisce risorse per 5,4 miliardi e definisce aumenti di spesa e sgravi fiscali per 12 miliardi». ancora: «Le recenti decisioni di politica di bilancio non frenano la dinamica della spesa».

la prima volta la spesa pubblica supera il 50 per cento del prodotto interno lordo. Insomma, a parere di chi si intende più di me di economia e di finanza, stiamo sperperando

un metodo di lavoro sul bilancio che si è rivelato disastroso, a partire dal 1978, quando fu introdotta la legge finanziaria. Citerò il ministro Padoa-Schioppa, che nel suo intervento del 3 ottobre scorso ha dichiarato: «È da augurarsi che non sia lontano il giorno in cui il disegno di legge di bilancio, che entra in Parlamento il primo giorno di ottobre, non abbia bisogno di una legge finanziaria che lo modifichi». Sottoscrivo queste parole. La finanziaria nacque, come certamente i colleghi sanno quanto me o anche meglio di me, per aggirare l'articolo 81 della Costituzione, voluto da Einaudi, che - come è noto - stabilisce che

Mi auguro, e lo annoto quasi a futura memoria, che si torni alla legge di bilancio semplice, il che significherebbe tornare alla normalità.

residente all'estero, ottenendo buoni risultati ma anche compiendo grandi rinunce. I senatori della circoscrizione Estero hanno dimostrato il loro senso di appartenenza e dello Stato, guardando all'interesse generale del Paese e non solo ai pur legittimi interessi della propria circoscrizione.

vivono, o meglio sopravvivono, al di sotto della soglia di povertà. Sono donne e uomini che hanno contribuito allo sviluppo dell'Italia del dopoguerra con le loro rimesse; donne e uomini che la vita non ha risparmiato e che oggi vivono in stato di indigenza. Il lavoro italiano nel mondo ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell'Italia contemporanea. Non tutti sono consapevoli che gli anni del miracolo economico italiano sono stati anche gli anni delle più grandi ondate di emigrazione e dei più grandi flussi di rimesse da parte degli emigranti. Nel dopoguerra, la più grande impresa italiana non è stata la FIAT, ma l'emigrazione, che, con le proprie rimesse, ha fatto vivere milioni di italiani e costruito migliaia e migliaia di case, per le quali oggi essi pagano le tasse. Presidente, cari colleghi e colleghe, in questi giorni abbiamo sentito parole offensive indirizzate ai senatori della circoscrizione Estero, in particolare, in Commissione bilancio, da parte del collega Polledri della Lega Nord. Voglio dire al senatore Polledri che le risorse per l'assistenza non sono destinate ai nipoti e alle zie dei senatori della circoscrizione Estero, ma a quelle donne e a quegli uomini che hanno contribuito allo sviluppo anche della Padania. Le sue parole non toccano e non raggiungono i senatori rappresentanti degli italiani nel mondo, ma offendono milioni di donne e uomini che, nel mondo, con il loro lavoro, con il loro attaccamento e il loro senso di appartenenza hanno fatto ben più che la loro parte per il progresso e l'ammodernamento dell'Italia. Quelle parole infangano solo chi le pronuncia! Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei far passare un solo messaggio e avere la capacità di far capire che la circoscrizione Estero e la presenza di parlamentari deputati dagli italiani all'estero sono più importanti per l'Italia che per gli italiani all'estero. È importante per l'Italia, per le sue esportazioni, per la presenza culturale economica e politica dell'Italia nel mondo, mondo, per l'ammodernamento e per la necessaria sprovincializzazione della politica italiana. Le risorse che la finanziaria destina alle Comunità italiane all'estero devono essere considerati come un investimento, e come un investimento con un ritorno veramente incalcolabile.

di soli sei Paesi europei, rendite pensionistiche per oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro. Questa cifra, poi, si può raddoppiare per la parte versata dalle Casse pensioni private, senza parlare dell'inestimabile indotto che gli italiani all'estero rappresentano per l'economia italiana sia per il turismo che per le esportazioni. Essi rappresentano la presenza viva del *made in Italy* che tanto successo riscuote all'estero. Signor Presidente, questo nel Senato della Repubblica, non interessi particolari o, peggio ancora, interessi personali un po' troppo presenti in quest'Aula. Concludo ringraziando i miei colleghi della circoscrizione Estero, i senatori Pollastri, Turano, Randazzo e Pallaro, che hanno svolto una riflessione e un lavoro collettivo, senza cercare di difendere interessi particolari e senza cercare una visibilità personale. Ringrazio anche la senatrice Rebuzzi, dell'opposizione, che ha condiviso con noi e il Governo un momento di riflessione comune. Noi non soffriamo della malattia, troppo diffusa in quest'Aula ed anche nella maggioranza, di cercare visibilità ad ogni costo, dimostrando così una grave assenza del senso di appartenenza, del senso dello Stato e della volontà di ricerca del bene comune. Noi questa malattia non l'abbiamo e spero che alcuni dei miei colleghi ne guariscano presto. Ringrazio anche il Governo, con il quale abbiamo ancora diversi confronti aperti e non risolti. Il principale è sicuramente la riforma della rete consolare, ma in questa fase della finanziaria abbiamo apprezzato la capacità di dialogo e lo spirito costruttivo dei sottosegretari Letta, Sartor e Grandi. Signor Presidente, colleghe e colleghi, per queste brevi e parziali considerazioni voteremo convinti questa finanziaria.

vivo ad Ascoli, in una città di provincia in cui le case del centro si vendono a 4.000 euro al metro quadro. Recentemente, un giornale locale ha sviluppato un'indagine conoscitiva sulle spese obbligate del bilancio di una famiglia media: moglie, marito e due figli. Considerando una casa di 100 metri quadri, un mutuo di 100.000 euro da estinguere in quindici anni, una trentina di prodotti ricorrenti nel carrello della spesa settimanale, le bollette di luce, acqua, gas e telefono, le tasse comunali, provinciali, regionali, le eventuali spese sanitarie e farmaceutiche, il costo della benzina e qualche spesetta varia, si arriva all'incredibile cifra di 1.755 euro al mese di costo della vita. Se tanto costano i beni di prima necessità in una città di provincia, immaginatevi nelle grandi metropoli. Un'altra domanda mi pongo e vi pongo. Se i livelli medi di stipendi e salari del nostro Paese sono di 1.000-1.200 euro al mese, una famiglia monoreddito arriva alla quarta settimana? Il tanto bistrattato Governo di centro-destra, con un sistema a scalare di deduzioni sulla base imponibile, aveva reso esenti da tasse oltre 13 milioni di redditi al di sotto dei 15.000 euro. Il Governo Prodi, nato «per il bene dell'Italia», ha cancellato le norme sul primo modulo fiscale. Sono state ripristinate le detrazioni fiscali, che hanno visto annullare con le addizionali regionali e comunali i modesti benefici riconosciuti con la precedente finanziaria dell'anno scorso, per i redditi al di sotto di 25.000 euro. I Comuni e le Regioni, però, non potevano fare diversamente! Con un raggiro contabile, infatti, avete svincolato il blocco delle addizionali per compensare i minori trasferimenti agli enti locali. Cosicché, a gennaio avete dato qualcosa con la mano dello Stato e ad aprile vi siete ripresi tutto con la mano degli enti locali. per i redditi superiori a 25.000 euro, avete preso sia a gennaio che ad aprile. Con i due "decreti Visco" e la finanziaria 2007, avete fatto una manovra da 38-40 miliardi di euro, più della metà dei quali consistente in nuove e maggiori tasse. Avete ingannato gli italiani dicendo che la manovra "di lacrime e sangue" era giustificata dal "buco" dei conti pubblici lasciato da Berlusconi. Non era vero niente. II disavanzo dello Stato nel 2006 è stato nei limiti concordati in sede europea. Già a novembre 2006 avevate registrato maggiori entrate, pari a 32 miliardi di euro, ma non le avete contabilizzate per non dimostrare che la manovra di risanamento era sbagliata perché infondata. Basta prendere i dati della relazione previsionale e programmatica del Governo Prodi: a settembre 2006 le entrate tributarie erano di 434,9 a settembre 2007 le entrate raggiungevano una cifra *record* di 474,5 miliardi di euro. In sedici mesi sono stati presi dalle tasche degli italiani, sia famiglie che imprese, ben 40 miliardi di euro. La metà di queste entrate sono state sono state ritenute strutturali ed hanno finanziato ben tre "tesoretti": uno a luglio di 7,4 miliardi di euro, uno a settembre di 6,3 miliardi di euro; uno con questa finanziaria, di 11 miliardi di euro. È da notare che un altro paio di miliardi sono in gestazione per finanziare, alla Camera, il raddoppio di 150 euro per gli incapienti previsto dal decreto-legge n.

Vantarsi che l'avanzo primario è aumentato al 2,5 per cento rispetto allo 0,6 per cento del 2005 del Governo Berlusconi, significa ignorare che tale risultato è stato ottenuto attraverso un aumento della pressione fiscale, che nel 2008 supererà il 43 Non solo noi dell'opposizione, ma il Fondo monetario internazionale, l'OCSE, la Commissione europea con il compagno Almunia, il governatore della Banca d'Italia Draghi, le più qualificate società di *rating*, valutano come superficiale o irresponsabile la politica di bilancio di questo Governo. Nessuno capisce come in un momento di espansione e di crescita dell'economia si possano destinare le maggiori risorse disponibili per spese clientelari ed elettoralistiche, anziché risanare il grande debito pubblico caricato sulle spalle delle future generazioni. La vostra irresponsabilità è ancora maggiore, perché sapete che l'euro è diventato una volta e mezza il dollaro e che il petrolio è arrivato a costare 90 dollari al barile: ciò significa per il 2008 e per gli anni seguenti più difficoltà di penetrazione nei mercati esteri, a causa dell'aumento del costo di produzione e di un aumento dei prezzi dei nostri prodotti, rispetto a quelli dell'area del dollaro. Questa politica da cicale si rivelerà disastrosa nel prossimo anno. Nel DPEF 2008-2011 del luglio scorso il Governo ha dichiarato solennemente che non avrebbe speso un euro senza aver tagliato un altrettanto euro di spesa inutile ed improduttiva: bugia, grande bugia! Avevate detto che avreste restituito agli italiani le maggiori entrate derivanti dal gettito tributario, invece non solo ve lo siete tenuto in gran parte per soddisfare la vostra base elettorale, ma quello che avete restituito è andato pure ai vostri elettori, dopo averlo prelevato a quelli che non vi avevano votato: anche qui bugiardi, ma anche pericolosi, perché non governate per l'Italia ma solo per i vostri amici e la finanziaria 2008 ne è l'ulteriore esempio. Abbiamo già fatto la lista della spesa parlando in occasione della conversione dei due decreti nn. 81 e 159. Penso sia giusto svolgere un'operazione verità chiarendo agli italiani quanta spesa clientelare contiene la finanziaria 2008. Avete previsto una maggiore spesa di circa 20 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi per spesa corrente e 11 miliardi per spesa in conto capitale. Tale nuova spesa corrente doveva essere finanziata, secondo il DPEF, tutta con altrettanti tagli di spesa; invece, la maggiore spesa la finanziate con l'extragettito tributario, che avreste dovuto restituire agli italiani, così come avevate scritto nel comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria 2007. Ma quale spesa finanziate? spesa finanziate? Gli incapienti? I disoccupati? I pensionati? La famiglia? La sicurezza? Le infrastrutture? Niente di tutto questo. Invece finanziate le aree confinanti, le minoranze slovene e le minoranze linguistiche, per tenervi buoni i voti al Senato del Gruppo degli autonomisti; un fondo per la presenza italiana presso le istituzioni europee e per gli italiani nel mondo, per tenervi buoni i senatori eletti all'estero; il contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani, le politiche migratone, il fondo contro la violenza alle donne e la cooperazione internazionale, tra cui la distruzione delle armi chimiche in Russia, prodotte dal vecchio regime comunista, per tenervi buona l'estrema sinistra comunista. Tutto questo, però, non è bastato, accontentava le forze politiche, ma non i singoli soggetti e i sottogruppi, che al Senato hanno un voto determinante. È successo così che, durante l'esame della finanziaria in 5a Commissione, la spesa corrente è aumentata per il solo 2008 di altri 2 miliardi di euro, mentre quella in conto capitale di 412 milioni. Nel triennio 2008-2010 la spesa complessiva è stata aumentata di circa 5,8 miliardi di euro, pari a 100 euro per ogni italiano. In questo elenco di spesa c'è di tutto: apicoltura, conservazione delle trincee della Prima guerra mondiale, i Giochi del Mediterraneo, le ferrovie venete, alcuni centri di alta specializzazione sanitaria, alcune aree verdi e la sicurezza idraulica di alcuni territori, alcune manifestazioni culturali e lirico-sinfoniche, il restauro di alcuni teatri e il Festival di di Puccini, il polo finanziario a Bolzano, i debiti residui delle Olimpiadi di Torino, il condono previdenziale per gli italiani all'estero che hanno percepito indebitamente le pensioni, il trasporto urbano, la ferrovia Pescara-Roma, i mondiali di nuoto, i contributi ad enti vari ed altre minutaglie. Come si vede, di alta politica o di interventi d'interesse nazionale non c'è niente. Noi dell'opposizione abbiamo cercato di incalzarvi su alcuni temi: famiglia, sicurezza, impresa, casa e giovani, infrastrutture. L'unico provvedimento del Governo che incideva sulla famiglia era la riduzione dell'ICI sulla prima casa. L'UDC, insieme alle opposizioni, ha presentato emendamenti con deduzioni decrescenti al crescere del reddito per i figli a carico, spese scolastiche, affitti, asili nido, spese sanitarie, congelamento estimi catastali, fondo rotativo per agevolare l'acquisto della prima casa. È stato questo confronto serrato che ha convinto la maggioranza ad approvare l'aumento della detrazione del 10 per cento sull'IRPEF per il caro mutui sulla prima casa; l'eliminazione del tetto di 50.000 euro di reddito per lo sconto ICI, che avrebbe penalizzato le famiglie monoreddito; la rimodulazione dell'assegno familiare per gli inabili; la deduzione, fino a 150 euro,

Dopo alcune esitazioni, un Governo diviso ci ha risposto con un provvedimento normativo che da solo non risolve il problema della criminalità. Se volete il sostegno dell'UDC sul "pacchetto sicurezza", le due misure devono marciare insieme. Le forze dell'ordine sono allo stremo: caserme sfrattate, volanti senza benzina e ferme per carenza di manutenzione; poliziotti, carabinieri, agenti di polizia penitenziaria senza straordinari e da anni con carriere bloccate; assunzioni insufficienti per garantire la rotazione dei pensionamenti (su 10.000 che se ne vanno, ne entrano solo 3.500). Di fronte a questo sfascio dello Stato, il centro-sinistra vara una norma per abolire la quota fissa di 10 euro sui *ticket* per prestazioni specialistiche ed ambulatoriali di contribuenti non esenti, ossia che non se la passano poi tanto male. Si tratta davvero di un pessimo esempio di senso dello Stato e di giustizia sociale, se si pensa che tale misura costerà alle future generazioni, in termini di debito pubblico, ben 834 milioni di euro. Sulle imprese, l'UDC, con l'opposizione, ha previsto una norma di salvaguardia per smascherare il raggiro della riduzione dell'IRES dal 33 al 27,5 Un altro caposaldo di questa finanziaria è la riduzione dei costi della politica. Su questo fronte il Governo è stato un campione di ipocrisia. Ha ridotto le spese per le indennità parlamentari, i costi del Parlamento, le indennità dei consiglieri regionali e gli amministratori locali, il funzionamento di Comuni, Province, comunità montane e società partecipate, per gli organi costituzionali

Signor Presidente,questa finanziaria è tutta una farsa. Spero di sì, ma non credo che questo Governo cada sulla finanziaria. Dini e i suoi amici e altri senatori comunisti dallo stomaco delicato digeriranno anche questo ennesimo pasto amaro. Occorre che la società civile sia più critica, meno conservatrice, più disposta a rischiare il cambiamento, alzi la testa e aiuti questa parte del Parlamento, che si oppone a questo degrado del Paese.

la strategia che la Sinistra Democratica ha messo in campo su questa finanziaria ha voluto avere come uno dei suoi punti principali l'attacco agli sprechi e ai costi impropri della politica,

dalle questioni che investivano, appunto, i vertici, il piano nobile, e non facendo volare gli stracci. Per questo, abbiamo guardato essenzialmente in tre direzioni: il Governo, la dotazione degli organi costituzionali, le maxiretribuzioni del settore pubblico.

riduce il numero dei Ministeri, si cancellano gli spacchettamenti (prima di Berlusconi e poi di Prodi), si introduce una novità, cioè il tetto complessivo di componenti a qualsivoglia titolo del Governo medesimo, fissato a 60.

In realtà, non poteva che farsi così. Non si può correttamente, dal punto di vista costituzionale, far cadere per legge un Governo. Non si può mettere un termine a tempo, con una norma legislativa ordinaria, perché è vero che il il Parlamento dispone della vita del Governo, ma attraverso uno strumento apposito che è l'articolo 94 della Costituzione. Per dare una spiegazione del perché non sarebbe stato costituzionalmente appropriato - lo dico per i giuristi e i colleghi costituzionalisti si sarebbe potuta determinare la possibilità che una norma di questo genere passasse in Aula con il voto per alzata di mano, annullando con ciò tutte le garanzie della personale e trasparente assunzione di responsabilità politica che, invece, l'articolo 94 impone con la procedura ivi prevista. Per questo motivo non si poteva che scrivere così quella norma. Si deve poi ovviamente auspicare sul piano politico che a quella norma il Governo e Governo e la maggioranza di centro-sinistra diano sollecita e tempestiva attuazione. Il secondo punto è stato la dotazione degli organi costituzionali.

Si è sentita subito qualche voce nel senso dell'inammissibilità, secondo alcuni, di questo emendamento, perché sarebbe stato lesivo dell'autonomia degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale cui si riferiva. È ben vero che si potrebbe, agendo sulla dotazione, incidere su tale autonomia, ma certo ciò non era vero per una regola generale nella sua portata, relativa a tutti gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e riferita ad una soglia più che ragionevole, come è l'incremento tenuto nel tetto dell'inflazione programmata. Quindi, a prima vista, *ictu oculi*, quell'emendamento non poteva dar luogo a nessuna lesione. lesione. Aggiungo che, ovunque, nell'esperienza moderna, gli appannaggi degli organi costituzionali vengono decisi dai Parlamenti. Del resto, anche da noi è così. Noi abbiamo nel bilancio una cifra che è riferita agli organi costituzionali e di rilievo che personalmente ritengo sciagurata - dell'inammissibilità, avremmo la curiosa conseguenza che a questo Parlamento sarebbe consentito soltanto sarebbe consentito soltanto autorizzare a piè di lista qualunque richiesta arrivasse dagli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Si tratta di una tesi palesemente inaccettabile e contrastante con l'esperienza costituzionale di tutti gli altri Paesi.

intervenire con regole prescrittive che nessuno può oggi più dubitare possano essere assunte. Abbiamo inteso stabilire - l'ho dichiarato esplicitamente in occasione del voto in Commissione bilancio - un precedente che chiarisse la titolarità del potere da parte di questo Parlamento e il fatto che gli impegni, da questo momento in poi, devono essere rispettati. Vengo alla norma sulle retribuzioni. Noi, già nella precedente finanziaria, avevamo introdotto un limite riferito alla alla retribuzione del primo Presidente della Corte di cassazione: per intenderci, una cifra intorno ai 270.000 euro all'anno. Questa regola, in realtà, fu resa largamente con la colpevole collaborazione del Governo, sia nella stesura del maxiemendamento, a tutti noto, sia nelle direttive adottate da Palazzo Chigi. Così quest'anno l'abbiamo con emendamento reintrodotta, con un carattere di maggior rigore: norma di generale applicazione, con previsione di deroghe assoggettate a limiti assai stringenti. Questa norma ha suscitato un allarme che, con ironia assolutamente consapevole, vorrei definire "sociale". Oggi sentiamo gli alti lamenti della RAI e perfino del Ministro (capisco che il Ministro difenda - lo dico in senso buono - i suoi *clientes*, mi sembra normale che accada così).

Io rispondo ai critici che i maxiemolumenti alla dirigenza RAI oggi in atto non hanno affatto garantito quella competitività. La TV di Stato è competitiva con Mediaset soltanto nei megastipendi. E, allora, se da quella parte, con qualche pesantezza, si dice che noi interveniamo in modo burocratico, da questa parte, con pari pesantezza, io dico che quei megastipendi sono un furto aggravato per le tasche dei contribuenti italiani. Personalmente, se la polemica dovesse continuare in questi termini, mi convertirò alla tesi della soppressione del canone, aprendo così la via alla possibilità che se poi i conti non sono in equilibrio, i libri della RAI si portano in tribunale. Se vogliamo aprire al mercato, facciamolo davvero, Ma la RAI è la punta di un *iceberg*. Noi abbiamo enti, autorità, società, organismi di ogni tipo, dirigenti, le cui le retribuzioni sono cresciute negli ultimi anni con un tasso di incremento non giustificato da più ampie responsabilità o funzioni, e talvolta con una crescita che ha addirittura coinciso con una diminuzione di responsabilità e funzioni. Una fascia ampia di retribuzioni d'oro di cui il Paese non sa, non è consapevole, anche se i contribuenti pagano di tasca propria. Proprio le maxiretribuzioni ci portano ad un altro punto che è qualificante per noi, e cioè quello degli emendamenti sui precari, perché le due cose si tengono insieme: precarietà e maxistipendi sono espressione del medesimo fenomeno che io ritengo degenerativo. La privatizzazione selvaggia della funzione pubblica, non sorretta da un solido orientamento politico e da una solida cultura istituzionale, ha prodotto questa degenerazione. Insieme precarietà e maxistipendi: in entrambi i casi aprendo la via ad estesi stessi fenomeni di clientelismo, di mala amministrazione e di mala politica. Da un lato, una troppa estesa precarietà, esternalizzazioni selvagge, funzioni strutturali affidate a personale assunto a tempo o con contratti di collaborazione precaria; dall'altro, megastipendi giustificati dal richiamo ad un mercato che in realtà non esiste. *Managers* che giustificano i propri emolumenti richiamando un privato che a quel prezzo non li assumerebbe mai. Così si è creata nel Paese una fascia ampia di retribuzioni d'oro accanto ad una fascia, di cui purtroppo il Paese è è duramente consapevole, di troppo ampia precarietà, nel quadro di degenerazioni di cui siamo altrettanto consapevoli. Non mi stanco di ripetere che Stella, Rizzo e Grillo sono effetto e non causa dell'ondata che oggi investe la politica e le istituzioni in questo Paese. Tutto questo non è un problema di pochi moralisti, diventa un problema del Paese. Lo dice il governatore Draghi quando sottolinea che esiste una questione salariale che deprime le prospettive di crescita complessiva. il presidente Morando quando richiamava il fatto che il confronto tra le parti sociali non ha corretto il dato dei salari troppo bassi. allora a Draghi e a Morando: non è forse causa di questo la troppo estesa precarietà che incide, appunto, sul confronto tra le parti sociali? E non è forse concausa il fatto che troppe risorse siano assorbite da un mondo di dirigenze e *management* pubblico che, almeno in parte, è parassitario e improduttivo, clientelare e super pagato? Concludo, signor Presidente, dicendo che questa è la mia opinione e questo è il senso dell'iniziativa della Sinistra Democratica. Non è il frutto di una visione pauperistica, repressiva o scioccamente moralistica, quanto piuttosto di una concezione diversa della cosa pubblicae della necessità, che noi riteniamo impellente, che l'equilibrio di questo Paese vada recuperato. mi attesto su ciò che oggi la finanziaria prevede. Ritengo politicamente decisivo che essa rimanga sostanzialmente nei termini in cui è, perché non difendo vantaggi di questo o quel territorio, di questa o quella corporazione o categoria, quanto piuttosto un'idea di giustizia